che all'inizio della sessione autunnale, pochi mesi fa, all'unanimità questa Assemblea aveva preso l'impegno di chiudere i lavori sui disegni di legge relativi al testamento biologico entro il 31 dicembre Grazie

Infatti, l'Assemblea è stata impegnata in questi mesi in modo molto consistente per la conversione di un numero straordinario e inusitato di decreti-legge e questo ha lasciato pochissimo spazio alla trattazione di altri argomenti, segnalarvi che la questione del testamento biologico è gravissima, riguarda un problema su cui giustamente l'opinione pubblica di questo Paese è molto sensibile e che

di trovarci di fronte alla circostanza che il Parlamento è chiamato o a convertire decreti-legge o a votare deleghe in bianco, generiche, al Governo,

il sistema e la funzionalità della pubblica amministrazione, parte già con questo limite (insieme a tutti gli altri provvedimenti che abbiamo approvato in questi mesi), non siamo messi nelle condizioni di svolgere un buon lavoro.

quale non produce la possibilità di un confronto adeguato al contenuto e al merito del provvedimento stesso. La prima contraddizione che rileviamo è che, da un lato, il Governo chiede una delega su questa materia,

che collega il provvedimento in esame alla legge finanziaria; dall'altro, ritiene poi non solo di prendersi un tempo lungo per l'esercizio della delega, ma di avere addirittura 24 mesi di tempo per poter intervenire con decreti delegati correttivi, integrativi o modificativi della normativa che intende introdurre. Se si tratta di materia strettamente connessa e collegata all'esercizio della funzione di Governo - e, nel caso di specie, alle manovre di bilancio e finanziarie, di cui il pubblico impiego è oggettivamente una parte importante - non si può poi pensare di prendersela comoda nell'esercizio della funzione normativa, perché ciò è incoerente, incongruente e, allo stesso tempo, contraddittorio.

Intanto, l'ambito d'applicazione di questa disciplina

della disciplina contenuta nella delega anche alla Presidenza del Consiglio. Le uniche funzioni specifiche, infatti, che non sono e non possono essere soggette alla disciplina organizzativa di questa delega, sono solo quelle che riguardano il disimpegno delle funzioni in materia di sicurezza, quindi legate ai cosiddetti servizi di prevenzione e sicurezza. L'ambito di applicazione di questa delega, invece, è ridotto. Ma è ridotto anche con riferimento ad un'altra area, perché non basta ritenere che queste norme possano costituire principi fondamentali ai fini della legislazione concorrente, della competenza concorrente tra Stato e Regioni. Lo Stato, signor Ministro, ha una competenza in materia di legislazione sugli enti locali, per cui credo sarebbe stata cosa buona e giusta estendere l'ambito di applicazione di questa disciplina anche, se non soprattutto, agli enti locali, che oggi disimpegnano una serie di funzioni importanti e sono, nel rapporto con il cittadino, il primo baluardo su cui inciampa il sistema della inefficienza dell'apparato pubblico. Ci saremmo aspettati, da questo punto di vista, un passo in avanti e una estensione degli effetti di questa normativa anche e soprattutto rispetto Non abbiamo gradito, ancorché sia stato apostrofato come un provvedimento demagogico,

se avessero avuto la forza di comprimere e tagliare la composizione quantitativa e qualitativa dei Gabinetti e degli Uffici dei Ministri e dei Sottosegretari, associando a questo anche una revisione sostanziale della disciplina in materia di *spoil**s system* e di selezione dei dirigenti.

- dobbiamo dare applicazione integrale all'articolo 97 della Costituzione, che afferma due principi fondamentali: il principio di imparzialità e quello di buon andamento della pubblica amministrazione. Il provvedimento in esame sotto il profilo dell'applicazione del principio del buon andamento introduce alcuni elementi di novità, ma sotto quello della garanzia della imparzialità della pubblica amministrazione incide solo per una parte, e cioè con quella parte della delega che interviene su alcune

della esecuzione e dell'indirizzo politico del Governo, ma anche a coloro i quali sono preposti a garantire che il settore della amministrazione di cui hanno la responsabilità sia efficiente. Ciò infatti non viene garantito in ragione del livello di fedeltà politica a questo o a quel Ministro, a questo o a quel Sottosegretario, a questo o quel partito, bensì dalla qualificazione professionale e dalla capacità di scelta di persone che siano all'altezza del compito e sappiano poi, a loro volta, selezionare

Noi abbiamo apprezzato e riteniamo fondamentale in questo provvedimento la decontrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego. Lo Stato e le amministrazioni pubbliche non svolgono una funzione imprenditoriale. L'interesse che tutelano non è privato,

La seconda considerazione è che non si attribuisce a questo soggetto il potere di determinare i criteri e le misure di valutazione del pubblico impiego, che in parte restano incardinate nella valutazione affidata alla contrattazione collettiva e in parte vengono attribuite alla valutazione del Governo.

una norma nefasta volta a riorganizzare il sistema di controllo svolto dalla Corte dei conti in quanto si attribuiscono competenze aggiuntive senza maggior personale e si snatura la funzione giurisdizionale vanificando il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

il Gruppo Italia dei Valori ha contribuito con impegno e serietà all'elaborazione in Commissione e in Aula di questo disegno di legge. Proprio per questa ragione ritiene di poter sottolineare con intensità molti elementi di critica in proposito. Il primo punto riguarda il contesto storico-parlamentare. Abbiamo affrontato questo disegno di legge già depurato di un fattore fondamentale, giacché presso la Camera dei deputati i tentativi volti ad individuare i criteri

che spiega la nostra insistenza rispetto agli emendamenti per tentare di limitare la potestà dei dirigenti. Sarebbe ingiusto che si attribuissero ai dirigenti potestà superiori proprio nel momento in cui si è impedito invece addirittura di ragionare soltanto sulla possibilità di individuare le loro responsabilità. Il secondo punto di critica (lo ha già trattato in maniera magistrale il collega D'Alia e quindi non ci ritornerò) riguarda i limiti della delega. Li richiamo soltanto perché non ha senso stare a ripetere una questione che è stata illustrata benissimo. I limiti della delega influiscono anche sul sul resto del provvedimento, perché insistono a rendere dubbio un quadro che potrebbe essere più preciso. Un terzo elemento di ragionamento critico su tale provvedimento di legge riguarda il dualismo, che è stato creato volontariamente o involontariamente nel corso dell'elaborazione tra istituzione di un'agenzia di valutazione e cancellazione della cosiddetta vicedirigenza. In astratto, l'idea di un'agenzia di valutazione è una questione ma questa dipende in parte dall'opacità della delega ed in parte è segnata da un costo francamente

qualche dubbio sulla possibilità che un'agenzia di questo tipo possa diventare un altro carrozzone di sottogoverno ci deve perlomeno sfiorare. La questione della vicedirigenza è controversa. Ieri il collega Passoni ha criticato con veemenza i nostri emendamenti in merito. comunque la si metta, si tratta di un provvedimento che nel 2002 aveva stanziato dei fondi nel bilancio dello Stato; questi fondi non sono stati attribuiti e devoluti dal sistema di contrattazione tra Governo e sindacati. Era una ragione di spesa già impegnata e non si riesce a capire perché se si ritiene fondamentale istituire un'agenzia di valutazione lo si debba a fare a spese di una ragione di spesa che era già stata impegnata. Il quinto punto di critica, forse in termini di principio il più veemente di tutti, riguarda la distorsione preoccupante cui è stata portata la Corte dei conti. Una legge nella legge, che istituisce tutto un processo di mutamento di questo ente di

è visibilmente in contrasto con la spirito che la legge vuole avere. Faccio soltanto l'esempio, che però è indicativo, della giustizia, dove 138 magistrati sono stati sottratti ai loro impieghi negli uffici di natura territoriale e convogliati negli Uffici di gabinetto, a fronte di una condizione che vede già il il fabbisogno territoriale della magistratura inferiore dell'8 per cento alle necessità. Insomma, mi accorgo di aver assommato, uno dietro l'altro, argomenti che porterebbero con coerenza a sostenere la possibilità di un voto contrario.

ad un'importante iniziativa di legge delega, che è stata esaminata ed arricchita dal lavoro proficuo svolto

È evidente che vi è una crisi di efficienza del lavoro pubblico, che da più parti è imputata anche alla sua diversa regolazione rispetto al lavoro privato. Durante gli ultimi anni si è tentato un avvicinamento ad un assetto di tipo privatistico e si è provveduto a disciplinare un nuovo assetto per la dirigenza pubblica. Si è dato particolare rilievo ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, potenziando anche gli istituti della mobilità e ridefinendo, a scopo di razionalizzazione, la disciplina dell'accesso al pubblico impiego. Tuttavia, rimangono ancora delle disomogeneità evidenti. Anche con questo disegno di legge delega si va nella direzione della convergenza del mercato del lavoro pubblico con quello del lavoro privato, stabilendo criteri direttivi relativi alla innovazione della disciplina sulla valutazione delle strutture e del personale della pubblica amministrazione. L'obiettivo è quello di innalzare gli *standard* qualitativi ed economici dell'attività amministrativa, attraverso gli strumenti della valorizzazione del merito e dell'incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa. È infatti importante abbandonare il residuo storico che identifica nell'impiegato pubblico il titolare di uno *status* (a volte anche di privilegi, a volte senza il necessario corrispettivo di servizi), approdando ad una condizione di lavoro attiva e responsabile. Quello che la nostra gente ci ha chiesto, sostenendoci con il proprio voto, e che ci chiede ogni giorno è di avere una pubblica amministrazione moderna ed efficiente, che dia risposte immediate e che non spenda inutilmente le nostre risorse. Il difetto di efficienza della macchina pubblica si ritraduce direttamente in riduzione della competitività complessiva del Paese, arrecando notevoli problemi a tutti i settori produttivi. Ed è a tal proposito che uno degli obiettivi qualificanti dell'azione di questo Governo è proprio il contrasto ai fenomeni di bassa produttività ed assenteismo. Questo obiettivo è stato già attuato tramite diverse misure che hanno portato a risultati importanti, in primo luogo il calo delle assenze dal luogo di lavoro per malattia. Infatti, come dichiarato in questi giorni dallo stesso Ministero, a novembre - se non mi sbaglio - le assenze per malattia sono calate del 41,4 rispetto allo stesso mese del 2007, con un evidente risparmio per il bilancio dello Stato. Quindi penso che l'azione del signor Ministro vada nel verso giusto. evidente che i provvedimenti adottati hanno indotto i dipendenti pubblici ad avere comportamenti più responsabili; un'ulteriore spinta verso la maggior efficienza del lavoro dei dipendenti pubblici verrà anche dall'approvazione di questo disegno di legge. Vi è l'esigenza di assicurare l'effettiva selezione concorsuale, sia per la progressione in carriera dei dipendenti pubblici, sia per il passaggio alla prima fascia dirigenziale. In particolare, è previsto che la valutazione positiva conseguita dal dipendente per un congruo arco temporale costituisca titolo rilevante per la progressione in carriera.

queste procedure prevedono il riconoscimento della rilevanza della residenza anche ai fini concorsuali e ciò costituisce uno dei fondamenti del programma della Lega Nord Padania. Nel merito, si riconosce che, conformemente al principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici, il principio della territorializzazione delle procedure concorsuali sia garantito mediante specifiche disposizioni del bando, anche con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili, o almeno non attuabili con identico risultato; ciò naturalmente senza voler discriminare nessuno. Un altro Un altro dei nostri obiettivi qualificanti in tema di lavoro pubblico riguarda l'adeguamento della contrattazione collettiva al diverso costo della vita nelle differenti aree del Paese.

In base alla Costituzione, il lavoratore ha diritto a una retribuzione sufficiente a garantire a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, ma l'eliminazione della scala mobile ha aumentato le disparità sociali. Per noi occorre dunque prevedere per il pubblico impiego la contrattazione collettiva su base territoriale

si richiedeva di attivare le procedure necessarie alla riforma del sistema della contrattazione nazionale del pubblico impiego e ad introdurre strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli territoriali di governo nella gestione della contrattazione collettiva. Ci auguriamo pertanto che tale fondamentale impegno politico possa essere a breve realizzato. In conclusione, e con questo auspicio al Governo, siamo convinti che dalla presente riforma possa nascere una nuova concezione di una pubblica amministrazione più efficiente e più vicina alle esigenze dei nostri cittadini.

colleghi, i senatori del Partito Democratico ritengono che sia indispensabile una riforma seria, profonda ed effettiva della pubblica amministrazione. Il Paese oggi paga un prezzo insopportabile in termini di competitività con gli altri Paesi per l'inefficienza della pubblica amministrazione; i cittadini, onorevoli colleghi, pagano un prezzo insopportabile in termini di qualità della vita di ogni giorno. Noi rivendichiamo il merito, negli anni in cui abbiamo guidato il governo del Paese, (con i ministri Cassese, Bassanini e Nicolais, solo per fare alcuni nomi) di avere provato a incidere in modo efficace sul ridisegno della pubblica amministrazione del nostro Paese. E, naturalmente, come fa chi opera scelte coraggiose, coraggiose, alcune le confermiamo ancora oggi, altre probabilmente andrebbero riviste. Oggi ci troviamo però nella condizione di scegliere le modalità con cui vogliamo intervenire. Signor Ministro, per mettere mano alla pubblica amministrazione del Paese ci sono due opzioni, una serie di provvedimenti, anzitutto legislativi, ma poi anche organizzativi e amministrativi seri, anche impopolari quando occorre, occorre, ma con un disegno di profonda modernizzazione; oppure si può fare la scelta che tante volte il Governo di cui lei fa parte preferisce, quella degli *spot*, qualche volta anche efficaci sul piano della comunicazione, ma che lasciano sostanzialmente inalterato il quadro normativo su cui si intende intervenire. Signor Ministro, voi in questo ambito avete iniziato scegliendo la strada sbagliata, la strada dello *spot*, quello della lotta ai fannulloni certamente è particolarmente efficace sul piano della comunicazione, e lei lo sa.

naturalmente considero la determinazione ed il coraggio con cui lei affronta alcune questioni un elemento a a cui guardare con attenzione. Ci è però sembrato, signor Ministro, che su questa vicenda lei sia stato mosso da un'ansia da consenso immediato, effimero, mentre non è così che si affronta una questione complessa e delicata come questa. Ci è sembrato che nell'avvio dei provvedimenti che lei ha posto in essere ci fosse una cultura prevalentemente, forse addirittura esclusivamente, punitiva. Questo, signor Ministro - voglio dirlo con grande chiarezza - non fa giustizia alle migliaia di dipendenti della pubblica amministrazione, di quella centrale come di quella locale, dai vigili del fuoco agli insegnanti, dai poliziotti a mille altre categorie, alle migliaia di persone che hanno

Ci è sembrato, cioè, che l'avvio dei provvedimenti che lei ha posto in essere, affrontando un problema vero e reale del Paese, fosse più sensibile agli approcci mediatici, ai problemi di comunicazione;

Era giusto inserire nel disegno di legge una maggiore efficacia nella valutazione del merito dei dipendenti pubblici,

quindi all'autorità amministrativa direttamente collegata con il Ministro, era sbagliata; così come non aveva senso escludere dal provvedimento in oggetto tutto il comparto degli enti locali e delle Regioni, che sono una componente essenziale della pubblica amministrazione in senso lato. Assolutamente inadeguate erano anche le norme che riguardavano il concetto di trasparenza, uno degli elementi essenziali se si vuole incidere efficacemente nel settore della pubblica amministrazione. Signor Presidente, il lavoro che è stato svolto nel Parlamento della Repubblica, in Senato in questa occasione, occasione, in una condizione di confronto aspro tra maggioranza e opposizione, tra Governo e minoranza, costituisce in qualche misura un'eccezione nel quadro politico in cui ci troviamo ad operare. Voglio dare atto pubblicamente, a nome dei miei colleghi, in particolare al Presidente della Commissione affari costituzionali, che è stato anche relatore del disegno di legge in oggetto, di aver operato con spirito di assoluta autonomia e senza pregiudizi, consentendo, anche con il lavoro del Comitato ristretto, che una parte significativa...

BIANCO *(PD)*. In un clima politico particolarmente infuocato e in una situazione delicata e difficile per il Paese, in Commissione affari costituzionali i colleghi di tutti i Gruppi hanno lavorato con grande passione, con grande competenza, facendo un lavoro parlamentare che giudico esemplare nella vicenda che stiamo affrontando. Voglio ringraziare pubblicamente coloro i quali hanno lavorato al Comitato ristretto, insieme con il relatore, e particolarmente - per quanto riguarda il nostro Gruppo - la collega Incostante, il collega Ichino e il collega Treu.

esame molte delle questioni importanti che in questa materia andavano affrontate. È stata costituita un'Autorità, una modalità di valutazione del merito nella pubblica amministrazione che si ispira a principi di autonomia e di indipendenza; non sarà la legge a regolare i rapporti sindacali all'interno della pubblica amministrazione, ma la normale dinamica contrattuale: quindi, non si fa un salto indietro di vent'anni in questa materia e si responsabilizzano i dirigenti.

in Aula) nella pubblica amministrazione, principio indispensabile per migliorare l'efficacia della sua organizzazione. Signor Presidente, intendiamo proseguire sulla strada della trasparenza e preannuncio che stiamo lavorando - è già pronto, il collega Ichino in particolare ci ha messo mano - su un disegno di legge particolarmente importante che riguarda la trasparenza e la pubblicità dei dei redditi e del patrimonio dei parlamentari, dei membri del Governo e di coloro i quali ricoprono cariche significative all'interno di enti pubblici di particolare rilievo.

siamo convinti che ci siano ancora margini di ambiguità e molto dipenderà da come saranno scritti i decreti legislativi di attuazione. Sappiamo che è un disegno di legge delega ovviamente occorre vigilare con grande attenzione affinché non si facciano nei decreti legislativi passi indietro. C'è un clima generale che continua a permanere all'interno del quadro politico su questa materia, signor Ministro, che non ci aiuta.

con le organizzazioni sindacali che certamente non aiutano e che destano grande preoccupazione. In particolare, sulla materia dell'assenteismo, un male che occorre combattere, si è scelta la strada di colpire con la scure

in considerazione del fatto che ieri in Aula sono stati approvati emendamenti che non hanno nulla a che vedere con lo spirito di questa riforma (mi riferisco, ad esempio, a quella brutta norma sui medici

di un Paese che vuole guardare avanti. Abbiamo lavorato in questo senso e lavoreremo con determinazione affinché il disegno riformatore prosegua. Per tali ragioni - ripeto

Attraverso il Comitato ristretto e la discussione svolta in Commissione, oltre che in Aula, riteniamo che il provvedimento sia stato ulteriormente migliorato e e segni un momento importante del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini. Il provvedimento va ad integrare, migliorare ed aumentare le prerogative

afferma che lei, ministro Brunetta, ha messo in essere uno *spot* quando ha parlato dei fannulloni. Lei, in modo icastico e molto comprensibile, ha sottoposto al Paese un problema che non sarebbe stato facile proporre in altro modo: ha parlato di fannulloni. I pochi che si sono sentiti fannulloni hanno immediatamente cercato di provvedere a esserlo meno; i tantissimi ottimi funzionari del nostro pubblico impiego si sono rallegrati di quella sua frase. Perché è così che si pongono i problemi, attraverso un'estrema semplificazione, di modo che poi l'attenzione si

Bisogna capire che la commissione deve essere esente da ogni tipo di condizionamento, per cui anche noi parlamentari dobbiamo autolimitarci su questo argomento. La Cassazione ha già detto che la raccomandazione non è penalmente perseguibile, ma forse sarebbe

e del senso della responsabilità. Tutti noi chiediamo questo, ma tanto più lo chiedono i lavoratori, i lavoratori, specialmente quelli del pubblico impiego. Se vogliamo - come vogliamo cambiare il Paese, dobbiamo renderlo più serio anche sotto questi profili, ripristinando il senso della gerarchia e della responsabilità. Come si lavorerà meglio quando i capi ufficio avranno la possibilità di seguire il lavoro dei loro subordinati, di indirizzarli e di correggere i loro errori!

come è stato detto, una legge punitiva. È una legge che finalmente porta avanti canoni di congruità che ci eravamo abituati ad aver perso. perso. È una legge, anche per il fatto che si sia realizzata con il concorso dell'opposizione, che sarà un faro per il prossimo legiferare. Lei ha messo in essere la

Queste cinque stelle polari sono quelle che riusciranno a cambiare il mondo del pubblico impiego. Mi auguro, ed in questo concordo con il collega collega D'Alia, che tali procedure vengano estese anche agli enti locali, perché è giusto. È negli enti locali che il cittadino ha il primo approccio per cercare di soddisfare le sue esigenze. l'approccio del cittadino, in questo caso nei confronti degli organismi statali, deve essere quello di chi va chi va per avere sorrisi e gratificazioni, tempi brevi e soddisfazione delle esigenze, attraverso, se è il caso, consigli; e non, come spesso accade, per trovare accade, per trovare soltanto difficoltà, paletti, problemi non risolti, rinvii ad altra giornata e poi ad altra giornata ancora. Quanto è importante quello che lei ha deciso, signor Ministro, e che il Parlamento le ha confermato, di mettere tutto su Internet! La grande trasparenza della pubblica amministrazione è poter vedere su uno schermo quel che accade di ogni pratica per capire come questa vada avanti, eventualmente per rivolgersi anche telematicamente alla pubblica amministrazione, onde dare un contributo per lo sveltimento della stessa. La sua idea di mettere a confronto costantemente i cittadini con le pubbliche amministrazioni è quello che noi cittadini vogliamo; sarà importantissimo il confronto. Così come sarà importantissima la fissazione degli standard qualitativi e di produttività e la possibilità di tutela

La conclusione obbligata, per i tempi che ho sforato anche se avrei avuto ancora tante cose da dire, è quindi estremamente positiva

la norma risulta ancora più snella; non c'è assolutamente motivo di pensare che si sia inserito in questo provvedimento un dato normativo estraneo:

alla logica del buon andamento gestionale. in quanto l'archivio della contrattazione, soprattutto di quella di secondo grado, è estremamente utile. È soprattutto utile in termini di trasparenza che tutta questa documentazione venga presentata al Parlamento e venga discussa in un convegno annuale, come previsto dalla norma. Complimenti dunque, signor Ministro. Prosegua in questa sua attività così svelta, così vivace, così competente e intelligente.

finestra"). Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indíco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 847 nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti», Dichiaro aperta la votazione.

Dopo l'illustrazione delle mozioni, ciascun Gruppo avrà a disposizione dieci minuti, comprensivi dei tempi della discussione e delle dichiarazioni di voto. Ha facoltà di parlare il senatore Rutelli per illustrare la mozione n. 67.

e ha conosciuto una notevole evoluzione... a nome dell'Assemblea. Colleghi, il senatore Rutelli deve illustrare la sua mozione e ha il diritto sacrosanto di farlo in un'Aula che lo ascolta o che quantomeno

dai cinque senatori che fanno parte del Comitato per la sicurezza della Repubblica. In quella sede, infatti, abbiamo ricevuto informazioni estremamente serie e preoccupanti su un fenomeno che sta assumendo una rilevanza strategica e non soltanto regionale, ovverosia la prateria che ha colpito decine

Grazie somalo e del prevalere drammatico delle fazioni, spesso armate, che si contendono il controllo di quel territorio e che nell'ultimo periodo di tempo hanno trasferito, per alcune organizzazioni territoriali criminali, i loro interessi economici sulla pirateria. Si tratta sorprendente per la sua dimensione, che s'immaginava appartenesse ad epoche del passato ma che invece ha un'incidenza enorme sul presente. Solo per fare una considerazione essenziale, signor Presidente, oggi un numero crescente di attività commerciali evita il Canale di Suez, con conseguenze economiche rilevantissime, in primo luogo per l'Egitto,

Quagliariello, Zanda, Passoni, Caforio, Compagna, Marcenaro e Carrara; successivamente il senatore Divina ed anche altri senatori del PdL hanno aggiunto documenti convergenti nella finalità della nostra iniziativa parlamentare, il cui scopo ha una fondamentale ragione: utilizzare gli ultimi giorni nei quali l'Italia siede al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Purtroppo, il trascorrere del tempo ha impedito che la mozione venisse trasmessa con istruzioni esplicite al Governo perché questo in seno al Consiglio di sicurezza si pronunciasse sulla materia in base ad un indirizzo parlamentare. L'intesa che in sede parlamentare e politica abbiamo stretto con il Governo, però, ha fatto sì che l'Italia, assieme assieme all'Unione europea e alle altre Nazioni interessate, abbia sostenuto una posizione assolutamente coerente con gli indirizzi di questi documenti parlamentari, che ora rapidamente riassumo. Il quadro di questa minaccia al largo del Corno d'Africa è in straordinaria e gravissima evoluzione e ci riguarda. Gli episodi di pirateria non sono isolati al largo delle coste somale. Nel corso del 2008, secondo l'Ufficio marittimo si sono verificati 92 attacchi a navi straniere a livello globale e attualmente sarebbero una quindicina le imbarcazioni sotto sequestro in acque territoriali somale e tra i 250 e i 300 i membri degli equipaggi tenuti in ostaggio. Solo nel mese di ottobre sono state attaccate 32 navi al largo dellaSomalia e, secondo dichiarazioni rese dal Ministro degli esteri del Kenya, sarebbero stati pagati oltre 150 milioni di dollari in riscatti di mercantili e altre imbarcazioni sequestrate negli ultimi mesi. Per intenderci: un ordine di grandezza di questo genere rappresenta più che le risorse di uno Stato. Stato. Si sta creando dunque, in alcuni territori della Somalia e con alcuni collegamenti che vanno oltre quei territori, un sistema di accumulazione di risorse che ha portato rapidamente a creare una infrastruttura, anche produttiva produttiva di mezzi in grado di recare attacchi ai mercantili in circolazione al largo di quelle coste e in un raggio di molte migliaia di miglia, perché vi sono stati sequestri al largo del Kenya, davanti a Mombasa, e altri in corrispondenza di Aden. Ci troviamo dunque di fronte ad una dinamica di una estrema gravità.

Secondo analisi internazionali solo nel porto di Eyl opererebbero oggi 5.000 persone collegate alle attività di pirateria, che investirebbero i proventi illeciti nella costruzione di nuove imbarcazioni. Secondo il Royal Institute of International Affairs di Londra il principale cantiere navale somalo, «Puntland Boat Manufactoring», riesce oggi a produrre un'imbarcazione di 18 metri munita di tre motori in meno di una giornata: siamo passati dai mitragliatori ai razzi, ai missili. Il 15 dicembre 2008 il Presidente somalo ha estromesso il Primo Ministro e l'intero Gabinetto di transizione, l'unico ad aver ottenuto un seppur fragile riconoscimento internazionale anche in seno all'Assemblea generale dell'ONU.

in particolare per garantire la consegna degli aiuti umanitari del programma alimentare mondiale e di altre agenzie del sistema ONU in direzione del Corno d'Africa e delle sue martoriate popolazioni. La missione della NATO originata da questa legittimazione internazionale ha visto la partecipazione di quattro navi militari dell'Alleanza atlantica sotto il comando dell'ammiraglio italiano Gumiero, cui va il nostro ringraziamento

della NATO che ho appena citato, ha preso il via la prima missione navale congiunta mai intrapresa dall'Unione europea, denominata «Eunavfor Atlanta». Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha approvato il 2 dicembre all'unanimità la risoluzione n. 1846, nella quale ha espresso forte sostegno a questa missione con comando operativo britannico. Come già previsto dalle diverse risoluzioni del Consiglio di sicurezza, i mezzi navali hanno il compito di garantire la sicurezza dei convogli umanitari in transito verso le coste somale e di scongiurare qualsiasi arrembaggio anche in acque territoriali della Somalia. Le regole di ingaggio consentono anche l'utilizzo della forza in caso di evidente minaccia o impellente pericolo. Una unità militare indiana ha affondato una nave di pirati circa un mese fa e si sono registrati altri interventi preventivi: un elicottero che si è levato in volo dal «Durand de la Penne», in almeno due circostanze ha impedito altri assalti ad altri convogli nell'area marittima. La missione attuale si compone di sei navi da guerra e tre aerei da ricognizione che devono sorvegliare una area che si estende per circa due milioni di chilometri quadrati, in cui rientra il Golfo di Aden. su proposta di diversi membri del Consiglio di sicurezza, appena l'altro ieri, 16 dicembre, il Consiglio stesso ha approvato all'unanimità una risoluzione, la 1851, che conferma l'impegno in Somalia, anche alla luce dell'intensificarsi degli atti criminali. Mentre stiamo parlando, colleghi, si sono registrati sequestri di altre tre navi. La mozione pone un punto politico rilevante: pur riconoscendo l'autorità esclusiva del Governo di transizione somalo sul territorio e sulle acque territoriali, così come previsto dai trattati internazionali, essa autorizza per un periodo di dodici mesi i mezzi militari coinvolti nella missione ad intraprendere qualsiasi operazione e ad utilizzare qualsiasi strumento, inclusa la forza militare, per smantellare le strutture logistiche dei gruppi di pirati, qualora (paragrafo 6 della risoluzione) il Governo somalo ne faccia esplicita richiesta al segretario generale dell'ONU. Concludo, signor Presidente. È evidente a tutti voi e a tutti noi che ci troviamo di fronte ad una delle conseguenze più drammatiche

le Nazioni Unite furono costrette a ritirarsi dalla Somalia. Quello fu uno dei più gravi fallimenti della comunità internazionale. Da allora ci siamo trovati di fronte ad un'esplosione di quel Paese. La nascita della pirateria con queste strutture logistiche a terra, fuori controllo (sono state sequestrate ed è tuttora sotto sequestro una nave con a bordo 100.000 tonnellate di petrolio, un'altra nave con a bordo decine di autoblindo e di mezzi militari, parte dei quali sarebbero già stati sequestrati e assunti dalle forze illegali della pirateria), ci pone di fronte ad un fenomeno di autentica rilevanza e di estrema gravità che è interesse della comunità internazionale mettere sotto controllo. È molto complesso e molte altre cose si dovrebbero dire, ma non voglio prendere altro tempo all'Assemblea che ringrazio per l'attenzione. I problemi, estremamente complessi, sono i seguenti. Cosa succede quando c'è un ingaggio? Cosa ne è dei pirati che vengono catturati? A quale autorità internazionale o nazionale riconosciuta vengono consegnati? A quale giurisdizione vengono affidati?

costruita sul campo, in un contesto così complesso e delicato. È molto importante, signor Presidente, che il Parlamento, in particolare, e per questa iniziativa, il Senato della Repubblica

possiamo definire un documento unitario, anche considerando che i testi depositati appena venti giorni fa sono superati dal drammatico svolgimento degli eventi cui ho fatto cenno in questa mia illustrazione. È un tema di grande importanza, che coinvolge il dovere di proteggere le popolazioni somale, di una regione in cui mancano gli elementi basilari per la sopravvivenza di centinaia di migliaia di persone e in cui non c'è Stato di diritto, non c'è affermazione di legalità e il flusso di risorse così consistente derivante dalla pirateria, è ragionevole valutare vada ad alimentare non solo organizzazioni criminali, ma anche attività terroristiche. Quindi, è un problema di enorme rilevanza rispetto al quale credo che il nostro Parlamento e l'Aula del Senato possano dare una risposta concorde ed efficace e una dimostrazione di coscienza e di concretezza particolarmente preziose. *(Applausi

a favorire tale intesa concedendo eventuali sospensioni della seduta o una dinamica dei lavori che consenta ai Gruppi di potersi separatamente riunire per arrivare ad un testo condiviso. Ha facoltà di parlare

Siamo convinti anche noi che, alla fine, dovremo riuscire a convergere su un documento unico; non sarà difficile, in quanto le varie mozioni mi sembra tendano tutte ad

Immediatamente è stata attivata una missione atlantica della NATO, anche perché vanno garantiti i traffici commerciali mercantili

di dotazioni straordinarie, quasi come un sistema navale organizzato statualmente. Quello che ci preoccupa sono le relazioni di polizia e di *intelligence* internazionale, che hanno ravvisato addirittura delle interferenze con il *network* jihadista e l'organizzazione di Al Qaeda, che probabilmente negli Stati falliti come la Somalia, ed in quelli in condizioni di sfascio istituzionale,

tuttavia ricordare un punto, che non è stato sottolineato da altri: la presenza militare in quel posto.

dal nostro Paese con l'ammiraglio Gumiero, che era al comando della missione atlantica in quella zona.

In questo momento capiamo qual è il problema: è più facile raccordarsi sotto l'egida europea, mentre può essere più difficile raccordarsi con russi, americani e addirittura indiani. Da parte nostra c'è l'esigenza di arrivare a delle regole di ingaggio comuni. Pur avendo fatto un grandissimo sforzo e una grandissima operazione,

un naviglio pirata è stata l'India, con la sua marina. Noi dobbiamo pensare che non è possibile partire con le mani legate nei confronti di un sistema di pirateria che non ha regole.

i pirati e per attaccarli eventualmente anche su basi di terra; altrimenti giocheremo sempre una partita impari, con una mano legata dietro la schiena,

dei pirati; sollevare in tutte le sedi internazionali competenti, soprattutto all'interno dell'Unione europea, un confronto sull'opportunità di estendere la lotta alla pirateria sul suolo della Somalia che ne ospita le basi;

Gravissimi sono i danni economici derivanti sia dai riscatti

ha sovrainteso alle operazioni di sicurezza del World Food Programme dell'ONU; nella seconda metà di dicembre la predetta forza navale della NATO è stata rilevata in area dalla prima missione navale militare dell'Unione europea, denominata «Atlanta», alla quale, per il momento, non prende parte l'Italia; a testimonianza della preoccupazione che la pirateria somala desta in seno alla comunità internazionale, per la minaccia che essa rappresenta per la sicurezza e per il regolare flusso degli aiuti umanitari destinati alle popolazioni dell'area,

in maniera assai incisiva i poteri delle forze impegnate nel contrasto alla pirateria. A questo punto, mi sembra improcrastinabile una nuova presa di coscienza del fenomeno da parte del nostro Paese e pertanto,

che siano adottate, in concorso con gli organismi internazionali e nel rigoroso rispetto del diritto internazionale, regole d'ingaggio adeguate all'implementazione delle misure di contrasto alla pirateria, ripristinando la piena utilizzabilità delle vie marittime, anche a scopo di assistenza umanitaria, come previsto dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU; ad adottare senza indugio provvedimenti diretti a consentire all'Italia di prendere parte alla missione navale dell'Unione europea A questo proposito, vorrei fare anche una precisazione che mi sembra utile nella nostra discussione, anche se non è attinente alle mozioni in oggetto.

soprattutto di fronte al fatto che vi è la volontà, da parte delle forze politiche in quest'Aula, di arrivare ad un testo comune. Il Governo non ha molto da aggiungere a tutto quello che è stato detto e concorda in linea di massima,

indicare cure per il sintomo è certamente un atteggiamento prezioso, però dimenticare la storia e la situazione della Somalia, secondo il Governo, sarebbe

Ringrazio il senatore Rutelli per aver ricordato che purtroppo la situazione del Governo transitorio somalo è peggiorata nell'ultima settimana, non è certamente migliorata. una seconda considerazione, peraltro già svolta dal senatore Cantoni. Siccome tutti noi stiamo operando ovviamente all'interno di un quadro di relazioni internazionali, di multilateralismo, sostanzialmente sotto un ombrello dato dall'ONU, voglio confermare che nel

vi è la possibilità, ovviamente da parte degli Stati membri, di adottare tutte le misure necessarie e appropriate in Somalia al fine di reprimere gli atti di pirateria e le e le rapine armate in mare a seguito di una richiesta del Governo federale transitorio somalo, che è stata interpretata - come credo tutti noi legittimamente interpretiamo - come disponibilità o possibilità, su richiesta del Governo transitorio somalo, di operare sui cieli della Somalia o addirittura sul territorio somalo. Questa interpretazione, che - ripeto - non si esclude, è però contraddetta da una notizia di questa notte secondo cui si è aperta una crisi, per il momento di relazioni, tra il Segretario generale dell'ONU e il Governo americano proprio sull'interpretazione circa la presenza di truppe di terra o dell'invio di truppe di terra sul territorio somalo onde porre in essere atti di contrasto alla pirateria. Quindi sarei più moderato nell'interpretare come possibili le operazioni a terra, usando perlomeno le parole che sono riportate nella Aggiungo un'altra notizia che può essere interessante: la Repubblica popolare cinese ha deciso l'invio di una propria forza navale nell'area.

Abbiamo avuto un rappresentante speciale italiano che ha operato quotidianamente, essendo presente a Nairobi, affinché si attivasse un processo politico-istituzionale di rafforzamento delle istituzioni somale.

altrimenti non si spiegherebbe - credo sia chiaro a tutti - come in alcuni porti del Puntland, che non l'ex Somaliland ma è una parte precisa da cui, tra l'altro, ha origine il presidente del Governo provvisorio Youssouf, c'è una situazione *in itinere* che va sempre più peggiorando. Le truppe etiopi si stanno ritirando e le bande degli Shabab, che sono in parte collegate alle Corti islamiche e quindi ad Al Qaeda (come è stato citato) rappresentano anche soltanto interessi di *business*, di traffico di droga e di armi e di altre questioni; come spesso accade, ormai la distinzione tra la parte ideologica e quella di criminalità organizzata è estremamente difficile.

Signor Presidente, affrontiamo oggi un tema di particolare attualità, che è stato oggetto di confronto nelle settimane passate sia alla Camera che al Senato in sede di discussione dei provvedimenti che il Governo ha inteso proporre per una riforma della scuola. Ci siamo fatti carico di portare all'attenzione dell'Assemblea del Senato il tema dell'integrazione dei minori stranieri nelle scuole perché credo che esso sia stato affrontato male e parzialmente anche in taluni dibattiti che hanno provocato alcuni pronunciamenti della Camera sulla stessa materia. Riteniamo che il fenomeno dell'immigrazione dei bambini e degli adolescenti stranieri sia crescente

Il secondo dato di riferimento è che il modo migliore per creare le condizioni per una integrazione degli stranieri e degli extracomunitari nel nostro Paese è proprio quello di partire dal mondo della scuola,

la presenza dei minori stranieri nel nostro Paese. Nel 2007 si stima, ad esempio, che nel nostro Paese siano nati 63.000 bambini di origine straniera. Si tratta cioè dell'11 per cento del totale dei nati in Italia nell'anno 2007 e quindi, tradotto in numeri più semplici, oltre un bambino su 10 risulterebbe nato da genitori con una cittadinanza diversa da quella italiana. Ancorché questo dato abbia tutta una serie di differenziazioni sotto il profilo territoriale, è estremamente significativo e va tenuto in considerazione. Se poi si guarda al dato complessivo dei minori stranieri nati o ricongiunti nel 2007 in Italia, ci rendiamo conto che, a fronte del totale fornitoci, ad esempio, dall'ISTAT, pari 767.060 minori,

Lo stesso ragionamento vale, signor Presidente, se guardiamo con attenzione ai dati che ci vengono forniti sulla presenza degli alunni di cittadinanza estera nelle scuole italiane. Nell'anno scolastico 2007-2008 si è visto che il numero degli studenti non italiani è salito del 14,4 per cento rispetto all'anno precedente, per raggiungere un dato complessivo

ed esclusivamente partendo dai minori, cioè partendo da coloro i quali vivono nel nostro Paese, sono arrivati nel nostro Paese, sono ricongiunti nel nostro Paese e che sono soggetti all'obbligo scolastico: quindi devono fare, secondo le leggi italiane, un percorso formativo che li metta nelle condizioni di poter apprezzare, conoscere e rispettare i nostri valori, la nostra cultura e la nostra Costituzione. Il modo migliore per fare questo non è quello di immaginare una separazione preliminare nell'accesso al percorso formativo, quello quello che viene esemplificativamente enunciato con l'istituzione delle classi ponte. Questo è un sistema sbagliato, perché segnala un'esigenza reale, cioè l'esigenza di fare in modo che l'offerta formativa e il sistema scolastico si adeguino alla crescente presenza della popolazione scolastica straniera. Ma al di là della segnalazione del problema, tende a dare una suggestione, anche di natura psicologica, sul modo di affrontarlo: facciamogli imparare l'italiano a parte; facciamogli imparare delle regolette di educazione civica, quasi che questo fosse il modo per consentire a bambini di cinque, sei, di considerarsi integrati; magari gli regaliamo pure un volumetto con la Costituzione e glielo facciamo leggere in maniera tale che siano nelle condizioni di concorrere con i loro coetanei italiani

di ripristinare le cosiddette classi aperte, che prevedano, senza eccessi, il raggruppamento di alunni bisognevoli di specifici interventi di insegnamento-apprendimento. Abbiamo bisogno di rafforzare i meccanismi previsti dal nostro ordinamento, che sono funzionali all'integrazione scolastica. Chiediamo scolastica. Chiediamo poi che il Governo si impegni a fornirci un quadro dettagliato ed aggiornato della situazione, individuando quali sono i punti di maggiore criticità. Abbiamo ascoltato e letto nei giorni scorsi che, ad esempio, in provincia di Bolzano è stata presentata

tentare di dare una risposta che faccia sì che vi siano le condizioni oggettive di integrazione all'interno delle classi e che il percorso formativo sia comune, ma anche adeguato alle diverse esigenze degli studenti, in ragione di ciò che questi sono in condizione di dare nel processo formativo al Governo di destinare risorse agli istituti e agli enti locali esposti su questo fronte. Abbiamo bisogno di intervenire rispetto a situazioni di criticità oggettive e non segnalando un problema generale senza avere il quadro del dato su cui

dei minori e degli studenti stranieri, con conseguente la necessità di intervenire con provvedimenti mirati a sostegno in quelle particolari zone. Nel Mezzogiorno d'Italia, viceversa, questo dato non ha una crescita esponenziale di particolare rilievo. rilievo. La nostra mozione, signor Presidente, tende a ripristinare un modo di concepire l'integrazione di studenti stranieri nel percorso e nel circuito scolastico all'insegna del buon senso, non dei manifesti ideologico né della necessità di invocare o evocare suggestioni.

culturali e formative diverse possano essere trattati allo stesso modo, però riteniamo che sia giusto che questo avvenga attraverso un percorso formativo unico in modo da creare le condizioni per un'integrazione le condizioni per un'integrazione che non sia solo scolastica, ma che diventi automaticamente integrazione sociale e culturale nel nostro Paese. Se si vuole realizzare un piccolo aspetto importante, e però strategico, di lungo periodo, delle politiche sull'immigrazione in questo Paese, bisogna partire da qui e bisogna farlo col piede giusto.

sollevano un problema reale. Nel nostro Paese sappiamo che gli immigrati regolari sono 2,5 milioni, e

abbiamo assistito ad un susseguirsi di strali da una parte e dall'altra:

dei Paesi, per così dire, meglio attrezzati a superare questa fase della crisi internazionale, debbano essere aperte a coloro i quali vogliono fare un salto positivo nella qualità della loro vita. Noi riteniamo che anche il concetto di cittadinanza debba essere posto all'esame del Parlamento. Questo non significa aprire indiscriminatamente le frontiere o snaturare il modo di vita, di pensiero e di cultura dell'Italia; significa, invece, migliorare insieme in un momento in cui la cultura multietnica è fondamentale fondamentale nella gran parte dei Paesi europei, e prima ancora negli Stati Uniti d'America. Siamo gelosi delle nostre culture, delle nostre tradizioni, delle nostre diversità, della nostra appartenenza allo Stato italiano e al nostro modo di pensare e di vivere, ma con altrettanta fermezza siamo contrari ad ogni forma discriminatoria all'interno del nostro Paese, ancora più grave se nei confronti di minori. ragione, tutti coloro i quali sono nell'obbligo scolastico devono essere integrati in ogni fase della loro vita e della loro giornata, non solo nella scuola nelle attività sportive e nelle attività di aggregazione sociale. Guai ad isolare i minori

Riteniamo che, come avviene per i nostri figli, che quando partecipano alle vacanze di studio all'estero vengono subito inseriti con altri, lo stesso debba accadere per i minori di culture diverse dalla nostra, senza classi separate e senza ghetti, ma con una forma di solidarismo culturale, fondamentale in una civiltà che si avvia ormai ad abbracciare e globalizzare la presenza delle Nazioni. Per questo chiediamo che il Governo, la maggioranza e tutte le forze parlamentari diano ascolto anche al messaggio del Santo Padre, che ha rivolto alle giovani generazioni di immigrati uno sguardo affettuoso, un abbraccio virtuale, ma reale, perché la tutela dei minori parte dalla migliore accoglienza. Per questo chiediamo che il Governo si criticità esistenti; a destinare, pur in questo quadro di difficoltà, maggiori risorse agli enti che, secondo la presente normativa, fanno fronte al problema dell'inserimento dei minori stranieri extracomunitari nella società italiana e a verificare se sussiste la necessità di modificare, come riteniamo, le norme attualmente in vigore, per raggiungere un progetto educativo nuovo, volto principalmente all'interscambiabilità delle culture e al pieno inserimento del minore all'interno di una società multietnica equilibrata. Chiedo di verificare se queste mozioni possano essere sapientemente sintetizzate in una unica, che possa trovare il consenso dell'intero Parlamento.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, vi sono tre mozioni, al nostro esame stamattina, che riguardano i minori immigrati nella scuola del nostro Paese. un tema intorno al quale si è acceso il dibattito, anche dopo la recente approvazione alla Camera dei deputati di una mozione della maggioranza, volta a introdurre le cosiddette cioè l'insegnamento della lingua italiana in modo separato e preordinato rispetto alle classi comuni. La mozione che qui intendo illustrare, per conto del Gruppo del Partito Democratico, affronta la questione della presenza dei minori immigrati nella scuola italiana per quello che essa effettivamente è, ossia una realtà nuova, di grande importanza per la costruzione della nuova società italiana. L'educazione e l'apprendimento dei minori immigrati insieme con i ragazzi italiani è l'anello fondamentale di ogni percorso di inserimento sociale. In questo quadro, l'integrazione linguistica e culturale è la chiave per dar vita ad un inestimabile capitale sociale, quello che si determina con l'integrazione. Questa è la nostra visione, culturale e politica, che vede nell'immigrazione - che segna potentemente il tempo attuale dell'Italia - un fattore strutturale, come hanno già detto i colleghi D'Alia e Belisario, che determinerà fortemente lo sviluppo e la coesione futuri del Paese. Per questo pensiamo ad un percorso organico d'integrazione, che fa dello stare insieme il criterio sostanziale e affida alla scuola, nella sua autonomia, la responsabilità di organizzare al meglio l'apprendimento, a partire da quello della lingua italiana. Sentiamo la responsabilità di questa sfida, perché qui è in gioco il futuro dell'Italia.

nell'anno passato era il 6,5 per cento), di 191 nazionalità diverse, distribuiti in ogni ordine e grado di scuola.

dopo la grande migrazione conosciuta nel Novecento verso l'estero da parte del nostro Paese e dal Sud al Nord negli anni Cinquanta. Se l'Italia oggi cresce e giunge, come ha ben rilevato Massimo Livi Bacci, a 60 milioni di abitanti è solo grazie all'immigrazione. In poche altre epoche della storia è stata così imponente la migrazione tra i continenti. Sappiamo che in taluni territori del nostro Paese, con classi in cui la presenza di alcuni immigrati supera il 40 per cento, si sta organizzando con equilibrio la loro iscrizione nelle scuole in modo da favorire una reale integrazione sulla base dei principi fondamentali,

e dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia. La pari dignità, il diritto all'istruzione, la non discriminazione, il riconoscimento della diversità come valore e arricchimento reciproco sono per noi la bussola per affrontare i problemi posti da questa novità. Queste sono le considerazioni, le premesse della nostra mozione. La mozione poi impegna il Governo ad un insieme di interventi coerenti e necessari, l'insegnamento della Costituzione e dei diritti umani, così che su questa base si costruisca il dialogo interculturale e interreligioso e una comune cultura civile e costituzionale dei ragazzi italiani e di quelli immigrati. Poi, si preveda che i minori siano ammessi in corso d'anno a scuola con le stesse regole degli alunni italiani; si garantisca la frequenza in classi miste per genere, etnia, lingua, religione perché la realtà è questa: le classi della scuola italiana sono eterogenee. Lì è la sfida culturale e sociale. Si deve potenziare l'attività didattica, i *curricula* in modo che l'apprendimento della lingua italiana possa avvenire con modalità flessibili per gruppi, laboratori, con corsi intensivi secondo l'organizzazione autonoma delle scuole, e sia favorita l'interculturalità. È dimostrato dalle esperienze e dalla ricerca che l'apprendimento della lingua italiana è più rapido se si vive insieme nello scambio. È riscontrato che vi è un anticipo di almeno sei mesi per il 60 per cento degli alunni che frequentano le classi comuni rispetto a quelli raggruppati in classi separate. Dobbiamo considerare che l'apprendimento linguistico è un processo più ampio della semplice conoscenza di un codice e ci conferma in questa impostazione la comparazione con l'esperienza degli altri Paesi, in particolare quelli con immigrazione storica. Venti anni fa in Francia le classi di ingresso, le classi d'*accueil*, separate per etnia hanno dato il risultato di un'altissima percentuale di bocciati. Occorre poi potenziare l'organico funzionale delle scuole, anche con mediatori culturali formati adeguatamente. Occorre dotare le scuole di testi e strumenti didattici adeguati che facilitino l'apprendimento della lingua italiana e delle lingue parificate - penso alle Regioni a statuto speciale - nonché l'interculturalità. Si debbono sostenere gli interventi degli enti locali che interagiscono con le istituzioni scolastiche. È necessario promuovere la partecipazione delle famiglie, soprattutto delle madri dei minori immigrati, delle associazioni degli immigrati, del volontariato, dell'associazionismo e si devono favorire i corsi per adulti, anche ai fini del conseguimento del titolo di studio. Insomma, una stagione di forte investimento sull'istruzione per l'immigrazione. per la promozione dell'educazione interculturale, nonché di programmi didattici multimediali e si devono anche potenziare gli istituti di cultura italiana all'estero per offrire corsi di lingua italiana sul posto. In sostanza, pensiamo che sia necessario prevenire il formarsi degli stereotipi, dei pregiudizi, dei fenomeni di razzismo e di xenofobia presenti e crescenti nel nostro Paese, favorendo il rispetto reciproco, lo scambio, l'integrazione nel solco della Costituzione perché è nella scuola che si mettono le basi di una futura convivenza civile serena e pacifica. Se i ragazzi vivono insieme a scuola, da grandi vivranno più facilmente insieme nella vita. Lingua e cultura si apprendono convivendo; l'integrazione si costruisce nello scambio: questi sono i pilastri fondamentali. Abbiamo esperienze molto interessanti: i ragazzi italiani sanno

Questa discussione parlamentare spero possa servire alla politica a non mettere ostacoli ulteriori sulla strada dell'incontro che la vita ha riservato, riserva e riserverà sempre di più ai ragazzi italiani ed ai ragazzi immigrati di oggi in questo nostro tempo di grandi cambiamenti. A mio parere occorrono pragmatismo, razionalità, idee fondamentali condivise ed una visione costruttiva, non negativa del futuro. Una visione che dirò semplicemente democratica, che non rinuncia mai a declinare nel futuro i principi fondamentali della libertà e dell'uguaglianza, l'eredità più grande della fatica dell'umanità. Questa è la sfida vera che sta di fronte a noi: non una Italia divisa, strutturata in una sorta di moderato e mediterraneo *apartheid* sociale, ci dice Livi Bacci, ma un'Italia integrata, con un'immigrazione di insediamento, di popolamento, di cittadinanza. Una nuova Italia, forte nelle sue radici, forte nella sua prospettiva.

Le mozioni presentate dai colleghi sottolineano un aspetto sicuramente importante. Credo che nessuno possa negare ragionevolmente l'importanza, anzi l'urgenza l'urgenza del fatto decisivo rappresentato dall'integrazione degli studenti di origine straniera nelle nostre scuole. Questo è un fatto assolutamente innegabile sul quale ci deve essere un forte impegno e non soltanto nel mondo della scuola. certo che questo punto sia all'attenzione del Governo, in particolare del Ministro, per questo non credo che siano particolarmente utili, se non a livello di

ad un'integrazione vera, che tenga conto della realtà e che non parta da presupposti ideologici. L'inserimento immediato e paritario a tutti i costi di persone che vengono da altri Paesi e in alcuni casi, non parlano la nostra lingua va affrontato secondo le necessità che si presentano di volta in volta. Non si può certamente ritenere che, comunque, ci debbano essere dei corsi di sostegno perché a volte arrivano nel nostro Paese persone parlano la nostra lingua oppure vi giungono così presto che l'apprendimento della nostra lingua avviene quasi in contemporanea con quello dei bambini italiani. Così come non si può pensare che un ragazzo straniero, magari cinese o arabo, che parla solo la lingua della sua famiglia possa facilmente inserirsi in una scuola media superiore. L'articolo 3 della Costituzione dice che la Repubblica rimuove gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della persona umana, ma in senso reale, non in senso psicologico; nel senso cioè che, se vi è qualche fattore che impedisce ad un cittadino di ottenere la piena parità con gli altri, la Repubblica deve agire per fare in modo che tale situazione venga superata e non far finta che non esista. io ho studiato anche all'estero, ma l'ho fatto dopo aver studiato a lungo la lingua del Paese in cui mi trovavo. Credo che se andassi a frequentare anche soltanto le scuole medie in Cina avrei qualche problema, pur avendo una preparazione culturale generale quantomeno discreta. allora che non si possa affrontare un argomento come questo in modo preconcetto e obbligando ad una scelta precostituita, indipendentemente dalle necessità. Occorre ricordare anche che compito proprio della scuola pubblica è quello di dare una base comune a tutti gli studenti che la frequentano, che siano italiani o di origine straniera.

per sé e anche per coloro che hanno deciso di votarli, grazie al fatto che hanno frequentato le scuole, in quanto

tutti cittadini di un Paese debbano conoscere le realtà del mondo che ci circonda; questo si è sempre studiato, anche quando l'immigrazione nel nostro Paese era praticamente nulla, ma ciò deve essere fatto per la conoscenza generale e non per sottolineare le per sottolineare le diversità. Credo che occorra dare una base comune, che deve essere quella di rendere la scuola un modo per salire socialmente, per inserirsi pienamente nella società; ciò non si raggiunge se l'inserimento deve

facendo carico alla scuola italiana di mantenere agli studenti anche la cultura dalla quale provengono. A questo ci penseranno loro, nella consapevolezza e nella cultura generale che dovrà loro dare la scuola.

le mozioni presentate dai colleghi e di cui oggi si discute esordiscono dichiarando che il fenomeno dell'immigrazione di bambini e adolescenti stranieri nel nostro Paese il loro inserimento nelle strutture scolastiche ha assunto dimensioni notevoli e tali da incidere in maniera rilevante sulla normale attività di insegnamento e apprendimento. La Lega Nord condivide appieno questo esordio e non ha mancato in molte sedi di entrare nel merito di quali siano le criticità rispetto all'espletamento della normale attività di insegnamento, apprendimento ed integrazione. Voglio qui ricordare alcune di tali criticità: difficoltà di apprendimento e, conseguentemente,

riescono a fornire loro un insegnamento adeguato e continuo della lingua italiana; difficoltà per le famiglie di tutti gli alunni che non vedono attuata per intero la programmazione annuale dell'attività concordata all'inizio dell'anno scolastico e coerente con le indicazioni nazionali, proprio perché la presenza di alunni che non conoscono l'italiano rallenta le attività scolastiche per tutti; realtà di plessi scolastici con percentuali di alunni stranieri che arrivano fino all'80 per cento e formazione, di recente, di singole classi di soli alunni stranieri, perché i dirigenti scolastici e gli enti locali non applicano la circolare ministeriale n. 110 del 2007, che prevede accordi di rete per favorire la distribuzione equa dell'utenza straniera sulle scuole dello stesso ordine presenti nel territorio. Infine, un progressivo abbandono da parte dell'utenza italiana della scuola pubblica verso la scuola privata e paritaria, anche perché non riconosce il multiculturalismo come valido mezzo all'integrazione. Sappiamo che gli elettori, non solo della Lega Nord, ma anche del centrosinistra, desiderano che i loro figli imparino ciò che prevedono le indicazioni nazionali e i curricoli regionali. Mi permetto di affermarlo perché noi siamo costantemente presenti sul territorio ed il territorio, sulla questione «multiculturalismo, sì o no», ha le idee sorprendentemente chiare, al di là dell'appartenenza politica. Vi assicuro, colleghi firmatari delle mozioni, che la scuola italiana non si è mai arrogata il privilegio di regolare i flussi migratori e mai lo farà: anzi, da sempre accoglie anche i figli dei clandestini. Ribadisco che educare al dialogo ed al rispetto per le diversità non significa rinnegare ciò che noi siamo, cioè relativizzare i valori della nostra cultura. Chi ha forti radici identitarie, chi ne è fiero e consapevole, è in grado di conoscere, rispettare ed integrare positivamente culture diverse. Chiedete corsi di formazione per docenti sulle tematiche dell'integrazione e della metodologia italiano Lingua 2: vi informo che, da anni, sono in atto corsi di formazione per i docenti docenti su queste tematiche in collaborazione con università, enti ed istituti di ricerca. Chiedete che le scuole a forte immigrazione ricevano più risorse da parte dello Stato: già lo Stato provvede in questo senso. Chiedete che si proceda all'equa distribuzione degli alunni stranieri sulle classi e sulle scuole: ebbene, nonostante le circolari ministeriali dei precedenti anni e, nonostante gli indirizzi che anche l'ex ministro Fioroni aveva indicato quali buone pratiche per l'integrazione degli alunni stranieri, per una sorta di ipocrisia buonista e di mancanza di coraggio da parte delle municipalità e dei dirigenti scolastici che tali pratiche dovevano applicare, aumentano nel Nord Italia le classi e le scuole con soli stranieri. Chiedete che ritornino le classi aperte o gruppi di alfabetizzazione: non sono mai state chiuse. Il problema è che funzionano per pochissime ore alla settimana e proprio per questo non riescono a colmare le lacune linguistiche degli alunni stranieri; anzi, vi informo che, fino a qualche anno fa, le classi aperte erano utilizzate per recuperare ed aiutare gli alunni italiani in difficoltà di apprendimento. Ora servono per aiutare gli alunni stranieri con difficoltà linguistiche. Chiedete che anche gli adulti stranieri possano avere corsi di lingua italiana presso le scuole elementari e medie, non sapendo che già esistono scuole per adulti pomeridiane e serali che offrono questo servizio. La mozione dei senatori del Partito Democratico chiede che i minori stranieri, oltre all'italiano, debbano anche imparare le lingue parificate delle Regioni a Statuto speciale, nonché la lingua inglese. Ma quante lingue straniere possono realmente imparare i minori stranieri, mantenendo l'attuale organizzazione scolastica, cioè quella indicata dall'articolo 45 del Regolamento di cui al DPR n. 394 del 1999, attraverso la quale, a fatica, accedono ad un livello sufficiente di conoscenza della lingua italiana? Chiedete che si arricchiscano i curricola obbligatori con contenuti relativi alle diverse culture, e sappiamo che in molte scuole sono presenti decine di culture diverse: così facendo togliete a tutti, italiani e stranieri, la possibilità di conoscere l'identità del nostro Paese, relativizzandone le radici culturali.

Per questo chiedo a tutti i colleghi senatori di riflettere su due semplici domande. Spogliandoci dell'ipocrisia e del buonismo superficiale, possiamo invece pensare ad una riorganizzazione scolastica più funzionale e pragmatica, al fine di aiutare gli alunni stranieri, che che non conoscono la lingua italiana, ad apprenderla in modo prioritario, veloce e ottimale, ottenendo così una reale integrazione ed un reale senso di appartenenza alla scuola italiana? Spogliandoci dei soliti luoghi comuni, è nostro dovere o meno tener conto che le famiglie italiane, insieme alle molte famiglie straniere che vogliono integrarsi, hanno il diritto di conoscere, apprezzare e fare propria la cultura del nostro Paese insieme alle tradizioni e ai linguaggi tipici dei diversi territori? La Lega Nord vi risponde che dobbiamo. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, il nostro Paese si è trovato negli ultimi vent'anni ad affrontare la crescita dei flussi migratori, un fenomeno che ha generato una situazione inedita per il nostro Paese. Di fronte ad una società diventata, di fatto, sempre più multiculturale e plurietnica e che, di conseguenza, ha visto le nostre scuole sempre più colorate con tante presenze di Paesi diversi nelle nostre classi, l'Italia ha già scelto la strada della piena integrazione di tutti nella scuola e dell'educazione interculturale come suo orizzonte culturale. L'Italia ha scelto, cioè, di valorizzare in pieno il significato del prefisso "inter", che rende bene l'idea di interazione, scambio, dialogo, apertura, reciprocità, solidarietà e, ad un tempo, rinforza il riconoscimento dell'identità culturale italiana, dei suoi fondamenti e dei suoi valori. La scuola ha scelto di dare senso al termine cultura, intendendola come riconoscimento dei sistemi di valori, dei modi di vita, delle tradizioni, delle credenze, dei diritti fondamentali degli esseri umani. Un riconoscimento in particolare è per i minori stranieri che, al pari di quelli italiani, sono anzitutto persone e, in quanto tali, titolari di diritti e doveri che prescindono dalla loro origine nazionale. Ne sono prova i numerosi provvedimenti normativi succedutisi dall'inizio degli anni Novanta ad oggi, che hanno gradualmente delineato in Italia una scuola delle cittadinanze, una scuola europea nel suo orizzonte, una scuola radicata nell'identità nazionale, una scuola capace di valorizzare le tante identità locali e, nel contempo, una scuola capace di far dialogare la molteplicità delle culture entro una cornice di valori condivisi. Questo è scritto nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del 2006. A fronte dell'impegno diffuso della scuola, delle buone pratiche, delle varie iniziative di accoglienza e di integrazione, permangono però molte questioni irrisolte nel processo d'integrazione. Di fronte ad una domanda d'istruzione e di formazione di giovani e di adulti immigrati di prima e di seconda generazione sempre più estesa, si evidenziano notevoli problemi e criticità e gli strumenti e i supporti attualmente disponibili appaiono insufficienti. Siamo di fronte a un'evoluzione del fenomeno immigrazione, un fenomeno diventato ormai un elemento costitutivo della nostra società e dell'identità della scuola italiana. La presenza di alunni stranieri è un dato strutturale riguardante l'intero sistema scolastico e la scuola riveste sempre di più un ruolo primario in quanto luogo dove, naturalmente, si educa al rispetto reciproco e alla convivenza democratica. Da qui sorge la necessità di aprire una riflessione profonda su questa nuova fase e sorge la necessità di ripensare l'azione educativa in cui avvengono lo scambio e il confronto fra culture. Si pone con urgenza l'esigenza di riprendere il dialogo sul tema dell'educazione interculturale e sul ruolo della scuola in questo particolare ambito di intervento. Diventano necessarie azioni che richiedono una rinnovata attenzione e un impegno organico del Governo, tali da determinare un'azione strutturale capace di sostenere l'intero sistema formativo nazionale. In ciò sta la continuità e l'esigenza di rideclinazione del compito assegnato dallo Stato nazionale alla scuola pubblica nazionale. Oggi, più che nel passato, il problema è quello di sostenere le istituzioni scolastiche, luogo naturale di accoglienza, di incontro, di confronto, di scambio, con strumenti e supporti efficaci per la piena integrazione degli immigrati, un sostegno nell'azione di riassumere la responsabilità, con scienza e coscienza, dell'incontro fra culture e di superare stereotipi e pregiudizi, per garantire, attraverso l'esercizio del diritto all'istruzione, piena cittadinanza. Si tratta di dare applicazione concreta ai princìpi della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, confermati nella Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989, ratificata dall'Italia nel 1991, principi che l'Italia ha fatto propri e che devono costituire un punto fermo per le politiche e gli interventi rivolti a bambini, ragazzi, adolescenti di ogni provenienza.

è una prospettiva che unisce la capacità di conoscere ed apprezzare le differenze e la ricerca della coesione sociale, in una nuova visione di cittadinanza plurale adatta al pluralismo attuale in cui si dia particolare attenzione a costruire la convergenza verso valori comuni radicati nella storia della nostra identità. In particolare, scegliere la prospettiva dell'educazione interculturale per la scuola significa non limitarsi a mere strategie di integrazione degli alunni immigrati, né a misure compensatorie di carattere speciale; significa piuttosto assumere la diversità come paradigma dell'identità stessa della scuola nel pluralismo, come occasione per aprire l'intero sistema a tutte le differenze e ciò sta nel DNA della nostra identità pedagogica nazionale. Significa riconoscere una valenza positiva alla socializzazione tra pari e al confronto quotidiano con la diversità, persistendo nella strada fino ad ora tracciata di integrare gli alunni di cittadinanza non italiana all'interno delle normali classi scolastiche. È una scelta che, come è stato di recente sottolineato in un documento di varie autorevolissime associazioni linguistiche, permette l'immersione nella nuova realtà linguistica e culturale e facilita il processo di acquisizione

L'acquisizione di una buona competenza nell'italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, è pertanto uno degli obiettivi prioritari nell'integrazione degli alunni stranieri in quanto rappresenta uno dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione sociale. pertanto, di porre una rinnovata attenzione all'apprendimento e allo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua, utile sia per comunicare che per apprendere nelle varie discipline e, quindi, per studiare. Per l'integrazione occorrono numerose azioni riconducibili a pratiche di accoglienza e di inserimento nella scuola, all'apprendimento dell'italiano come seconda lingua, alla valorizzazione del plurilinguismo, alla relazione con le famiglie straniere e all'orientamento. occorrono linee di intervento circa le relazioni a scuola e nel tempo extrascolastico, le discriminazioni e i pregiudizi, le prospettive interculturali nei saperi e nelle competenze. in modo molto approfondito nelle indicazioni per il *curriculum* della scuola di primo ciclo. Sono quindi necessarie linee di intervento che hanno a che fare con l'autonomia e con le reti tra istituzioni scolastiche, la società civile e, soprattutto, il territorio, a partire a partire dalla consapevolezza che l'integrazione si costruisce insieme, a scuola e fuori dalla scuola. Ed è proprio su tali azioni e linee d'intervento che oggi chiamiamo il Governo a confrontarsi e ad impegnarsi.

sia come appartenente alla 7a Commissione, sia come insegnante per attività professionale. I documenti che ci troviamo ad esaminare si muovono, a mio giudizio, secondo una filosofia che non solo non condivido, ma che non corrisponde nemmeno alla situazione che ho potuto sperimentare in forma diretta. della mozione n. 42: «le cronache quotidiane segnalano l'insorgenza di forme, più o meno palesi, di un certo razzismo che spesso determinano un sentimento di ostilità, di repulsione e che, a volte, generano violenze vere e proprie». Lo stesso concetto è ripreso nella mozione n. 69, laddove si legge: «le cronache di questi ultimi mesi indicano chiaramente un aumento di episodi di intolleranza e o razzismo, che spesso sfociano in atti di violenza vera e propria, soprattutto nei confronti di minori stranieri». Questo quadro, a mio giudizio, non è assolutamente veritiero; la realtà ci porta invece una situazione completamente diversa, con bande di giovani magrebini, di giovani albanesi, per non aprire il ragionamento ai nomadi, che meriterebbero un approfondimento a parte. In molti istituti, in molte realtà urbane si è creato un clima di intimidazione, di violenza, di cui sono vittime gli studenti italiani. Questa è la realtà così come viene conosciuta direttamente nelle nostre città. Un secondo passaggio riguarda la cosiddetta ottica dell'interscambiabilità delle culture. Credo che le culture siano legittimamente diverse, che questo sia un arricchimento per la comunità internazionale, ma penso che sia un dovere per tutti noi salvaguardare quel patrimonio quel patrimonio del sistema educativo e formativo italiano che poggia su valori che sono stati trasmessi generazione dopo generazione, di padre in figlio, sono sedimentati nella nostra comunità e rappresentano un elemento identificativo assolutamente irrinunciabile.

tale preoccupazione perché è fonte di un'effettiva discriminazione sociale. Chi vive in quartieri periferici, in quartieri marginali delle città, ha due opzioni: o un livello di apprendimento incompleto e limitato o il trasferimento in un'altra scuola o in un istituto privato. Questa è la situazione nella quale si trovano a scegliere alcune famiglie ed è effettivamente necessario prendere i provvedimenti del caso. è poi la questione delle cosiddette classi aperte; la formulazione è generica perché non si distinguono i livelli. È chiaro che nella scuola elementare serve un determinato tipo di sensibilità, nelle scuole medie inferiori e superiori il quadro è diverso. Ho vissuto un'esperienza alle scuole superiori; nella Provincia di Trento, governata dal centrosinistra, è arrivata una circolare della sovrintendenza che invitava ad inserire gli alunni stranieri nella classe corrispondente per età. immigrazione, appena arrivato ad esempio dal Ghana, veniva inserito a 16 anni in terza superiore, laddove per arrivare in terza superiore lo studente italiano doveva avere il diploma di licenza media inferiore, doveva superare una prima classe nella quale la selezione era intorno al 25 per cento, doveva arrivare in seconda e accedere successivamente alla terza. Si andava oltre come previsioni, nel senso che per quello stesso ragazzo veniva attivato un comitato di accoglienza, nonché una specifica commissione ricorso ad un mediatore culturale e, se serviva, ad un facilitatore linguistico. Alla fine dell'anno - queste erano le indicazioni - se il mediatore culturale sosteneva che il ragazzo aveva avuto dei progressi (e questa era la sua funzione, quindi i giudizi andavano in questo senso), il ragazzo era promosso, mentre lo studente italiano doveva avere comunque la sufficienza nelle diverse discipline. Se poi il mediatore culturale, negando l'efficacia del proprio lavoro, avesse scritto nella relazione che il ragazzo non aveva manifestato progressi di sorta, veniva promosso comunque con un progetto che veniva trasmesso per l'anno successivo. successivo. Scelte di questo genere non solo alimentano il razzismo perché creano oggettiva discriminazione nei confronti degli studenti italiani, ma non rappresentano neanche una soluzione al

Le tematiche relative all'integrazione degli alunni stranieri sono state già esaminate nelle sedute dell'Assemblea della Camera del 9 e 14 ottobre ultimo scorso, in occasione della discussione di varie mozioni al riguardo presentate

Si premette sinteticamente il quadro normativo di riferimento. Come è noto, in applicazione dell'articolo 10 della Costituzione, sono state recepite nell'ordinamento italiano le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute ed in particolare quelle puntualmente richiamate nelle premesse della mozione del senatore Giambrone, ivi comprese la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la Convenzione sui diritti dell'infanzia, richiamate pure nelle premesse della mozione della senatrice Soliani. Per quanto riguarda la condizione giuridica dello straniero, le norme regolatrici sono contenute nella legge sull'immigrazione 6 marzo 1998,

indipendentemente dalla regolarità della loro posizione in ordine al permesso di soggiorno, e pone attenzione sugli aspetti organizzativi della scuola, sull'insegnamento dell'italiano come seconda lingua, sul mantenimento della lingua e cultura di origine, sulla formazione dei docenti e sull'integrazione sociale. In attuazione della suddetta normativa sono state a suo tempo diramate dal Ministero, con circolare n. 24 del 1° marzo 2006, le «Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri». Va pure ricordato, per completezza, il documento «La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri», presentato nell'ottobre 2007 ed elaborato dall'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale, interculturale, istituito presso il Ministero dalla precedente gestione con decreto del 6 dicembre 2006. Passiamo, quindi, all'esame degli impegni previsti dal dispositivo delle mozioni in discussione. Considerato che le mozioni dei senatori D'Alia e Giambrone presentano alcuni profili comuni, procederò innanzi tutto all'esame dei dispositivi di queste, per poi procedere all'esame dei numerosi punti della mozione Soliani. identico impegno previsto dalla mozione D'Alia e dalla mozione Giambrone, viene chiesto al Governo di fornire un quadro dettagliato ed aggiornato della situazione, indicando i punti di maggiore criticità. A tal proposito, si fa presente che i dati analitici della situazione sono contenuti nella pubblicazione del luglio 2008 su «Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano», relativa all'anno scolastico 2007-2008, curata dal Servizio statistico del Ministero, reperibile anche nel sito Internet del Ministero medesimo. Per l'anno scolastico 2008-2009 la rilevazione è in corso. Nel rimandare, per il dettaglio, a tale pubblicazione, si evidenzia che dalla suddetta indagine risulta che in questi ultimi anni il cambiamento nella scuola italiana è stato rapidissimo. Dai 50.000 alunni stranieri dell'anno 1995-1996 si è passati agli oltre 500.000 nel 2006-2007 e a 574.133 unità nel 2007-2008, che rappresentano il 6,4 per cento del totale degli alunni. Alla popolazione straniera residente va anche aggiunta quella irregolare, la cui componente in età scolare ha pieno diritto e dovere di partecipare al sistema scolastico italiano, come previsto 394 del 1999, all'articolo 45. Le scuole primarie e secondarie di primo grado accolgono il maggior numero di allievi di origine straniera, che rappresentano rispettivamente, in percentuale, il 7,7 per cento e il 7,3 per cento dell'intera popolazione scolastica. L'analisi degli iscritti stranieri alla scuola secondaria di secondo grado per tipo di scuola fa emergere la tendenza verso gli istituti professionali e gli istituti tecnici, dove rappresentano, rispettivamente, l'8,7 per cento e il 4,8 per cento del totale degli studenti. Particolarmente significativa, per le necessarie riflessioni in ordine alle connesse difficoltà organizzative e didattiche, risulta la constatazione della presenza di alunni provenienti da oltre 150 diversi Emerge, inoltre, la mancanza di regolarità scolastica tra gli studenti con cittadinanza non italiana e ciò rappresenta un dato particolarmente allarmante, dovuto sia a difficoltà legate alla conoscenza della lingua italiana, che a problemi di integrazione sociale. In media, il 42,5 per cento di alunni stranieri non è in regola con gli studi e il crescere dell'età aumenta il loro disagio scolastico. Lo studio sul fenomeno delle ripetenze comprova il quadro già riscontrato in base all'età: per tutti gli ordini di scuola e per tutti gli anni di corso la percentuale di ripetenti stranieri è superiore a quella degli italiani. L'osservazione a livello territoriale evidenzia la disomogeneità della presenza di alunni stranieri nelle varie Regioni italiane. L'incidenza degli alunni con cittadinanza non italiana è particolarmente significativa in Emilia-Romagna, Umbria, Lombardia e Veneto, dove rappresentano più del 10 per cento della popolazione scolastica regionale. Va sottolineato che, in base al *Report* del Ministero riferito all'anno scolastico 2006-2007, sono 888 le le istituzioni scolastiche che superano il 20 per cento di presenze di alunni stranieri, ma tra queste ve ne sono 89 che superano il 40 per cento. La maggior parte di esse è concentrata nelle Regioni del Nord: Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte. Tra le Province con il maggior numero di scuole con significativa concentrazione troviamo Milano, Torino, Bolzano, Roma e Brescia, Le situazioni di criticità derivanti dalla crescente dimensione del fenomeno risultano particolarmente acute nelle aree in cui è più alta la concentrazione di alunni stranieri; si registrano, infatti, percentuali elevate al punto che il numero di alunni di diversa nazionalità e/o etnia presenti in classe in taluni casi supera persino il numero di alunni italiani, determinando notevolissime difficoltà organizzative che si riflettono negativamente sull'efficacia dell'inserimento degli alunni stranieri con rallentamento del processo di insegnamento-apprendimento per tutti, sia stranieri che italiani. Non v'è dubbio che la scuola ha un ruolo prioritario nel processo di integrazione in quanto sede privilegiata nella quale può opportunamente realizzarsi l'integrazione tra culture, il libero scambio e il confronto delle idee, la *par condicio* tra i soggetti che la frequentano, la crescita umana, civile e culturale delle nuove generazioni, al di là delle differenti etnie, nel rispetto dell'articolo 3 della Costituzione. Per assolvere a tali compiti, la cui complessità e delicatezza sono testimoniate dalla pluralità di modelli di integrazione adottati dai vari Paesi, la scuola deve dotarsi di strumenti adeguati, che consentano di far fronte alle nuove e molteplici esigenze attraverso servizi educativi, figure professionali, come i mediatori culturali, e metodologie idonee allo scopo. Particolarmente importante a tal fine è la collaborazione tra le istituzioni scolastiche, da un lato, e le Regioni e gli enti locali, dall'altro, che sono chiamati a collaborare al processo di integrazione degli alunni stranieri. È di tutta evidenza che lo strumento indispensabile, anche se non l'unico, per una effettiva integrazione degli alunni stranieri è quello della conoscenza della lingua italiana. Spesso i ragazzi stranieri sono inseriti nelle classi indipendentemente dal livello di conoscenza della lingua italiana ponendo problemi di tipo didattico ed organizzativo, con la conseguenza che risulta rallentato per tutti, sia italiani che stranieri, il processo di insegnamento-apprendimento. La primaria esigenza è quindi quella di insegnare la lingua italiana e la Costituzione della Repubblica, al fine di integrare pienamente nelle classi gli alunni stranieri che, pur con competenze proprie, risultano penalizzati dalla barriera linguistica. L'alfabetizzazione letteraria deve procedere di pari passo con quella civile, sia per i figli degli stranieri, che devono apprendere le regole della comunità italiana, sia per i giovani italiani. Ciò rilevato, alla luce delle criticità emerse e della crescente presenza di alunni stranieri nelle classi, il Governo, in riferimento al secondo ed identico punto del dispositivo della mozione Giambrone e della mozione D'Alia ed in riferimento, altresì, al terzo ed ultimo punto della mozione Giambrone, intende valutare il fenomeno ed apprestare più incisivi interventi per favorire un effettivo e proficuo inserimento degli alunni stranieri. Per ciò che concerne specificamente le risorse finanziarie, si ricorda che specifici finanziamenti in proposito sono previsti nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, in particolare all'articolo 9, che reca «Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio e a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica», e all'articolo 69, concernente la «Formazione per il personale delle scuole in aree a rischio o a forte processo immigratorio o frequentate da nomadi». Inoltre, per tali finalità la direttiva ministeriale del 6 agosto 2008, n. 69, relativa alla ripartizione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa, destina tre milioni di euro a progetti promossi e realizzati a livello nazionale per le attività di formazione e aggiornamento del personale della scuola nonché otto di euro per la prosecuzione di progetti riferiti, tra l'altro, anche all'insegnamento della lingua italiana. Passando agli ulteriori punti del dispositivo della mozione del senatore D'Alia, si fa presente quanto segue. Per quel che concerne il quarto e il quinto punto, va rilevato che sono già previste sia la diffusione delle buone pratiche che l'equilibrata distribuzione degli studenti stranieri. Altrettanto dicasi per il sesto punto, relativo al coinvolgimento delle famiglie nell'apprendimento della lingua italiana, che va incontro all'indirizzo ministeriale di fare dell'alfabetizzazione linguistica e civile la chiave di volta delle politiche inclusive. In proposito, si ricorda che la menzionata direttiva n. 69 del 6 agosto 2008 destina 20 milioni di euro per le iniziative, promosse a livello nazionale, dirette a realizzare, tra l'altro, anche l'accoglienza e il sostegno degli studenti con famiglie straniere. Quanto al settimo punto, relativo al ripristino delle classi aperte, si ricorda che esiste già il programma denominato «Scuole aperte». Con riguardo all'ottavo punto, relativo ai *curricula*, tenuto conto della ripartizione delle competenze tra lo Stato e le autonomie scolastiche, eventuali scelte di contenuto che abbiano a riferimento le varietà culturali sono riservate ai POF (Progetti di offerta formativa) delle stesse autonomie scolastiche, nell'ambito della quota a loro riservata, e alla libertà di insegnamento, ferme restando le Indicazioni nazionali, che rappresentano il comune denominatore dell'unitarietà della scuola italiana tante volte evocata. Per ciò che concerne, infine, l'ultimo punto della mozione D'Alia, si osserva che la differenziazione dei programmi appare incompatibile con l'esigenza di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi di tutti gli studenti. Quanto sopra per quel che concerne la mozione D'Alia e la mozione Giambrone. Venendo agli impegni previsti dal dispositivo della mozione Soliani, si fa presente quanto segue. si osserva che, invero, il Governo è già fattivamente impegnato nell'attuazione delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, recepite nell'ordinamento nazionale, in applicazione dell'articolo 10 della Costituzione, ed in specie della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e della Convenzione sui diritti dell'infanzia; ciò, secondo quanto detta l'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione. Circa il secondo punto, si ricorda che l'Assemblea della Camera, nella seduta del 14 ottobre ultimo scorso, ha approvato la mozione dell'onorevole Cota ed altri 1-00033 (Ulteriore nuova formulazione) la quale, al fine di un razionale ed agevole inserimento degli studenti stranieri, impegna il Governo a non consentire in ogni caso ingressi nelle classi ordinarie oltre il 31 dicembre di ciascun anno. è indubitabile che la frequenza dei cicli di istruzione avviene nelle classi ordinarie nell'ambito di classi miste per genere, etnia, lingua, religione, nel rispetto dell'articolo 3 della Costituzione. Relativamente al quinto punto, si rimanda a quanto già osservato circa l'ottavo punto del dispositivo della mozione del senatore Giambrone, riferito ai *curricula*. In merito al sesto punto, è indubbio che il ricorso ai mediatori culturali e linguistici agevola l'inserimento nel contesto scolastico degli alunni di altri Paesi e consente a quelli italiani di stabilire con i coetanei stranieri rapporti improntati improntati al reciproco rispetto, favorendo così il processo di integrazione e lo sviluppo nei giovani di una mentalità aperta e flessibile. A tal proposito va sottolineato che gli enti locali sono chiamati a collaborare al processo di integrazione degli alunni stranieri, spettando loro di mettere a disposizione delle scuole dette figure professionali. In ordine al settimo punto, concernente i libri di testo e gli strumenti didattici, nel richiamare quanto precedentemente detto circa i *curricula*, si ricorda che la materia dei libri di testo e degli strumenti didattici, essendo riconducibile alla libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente, è dall'ordinamento giuridico rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche; in particolare, è rimessa al collegio dei docenti che, avendo potere deliberante in materia di funzionamento didattico nel rispetto della libertà di insegnamento, garantita a ciascun docente, provvede all'adozione dei libri di testo e alla scelta dei sussidi didattici. Con riferimento all'ottavo, nono e decimo punto del dispositivo, si ribadisce che la direttiva ministeriale 6 agosto 2008, n. 69, relativa alla ripartizione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa, destina tre milioni di euro a progetti promossi e realizzati a livello nazionale per le attività di formazione e aggiornamento del personale della scuola nonché otto milioni di euro per la prosecuzione di progetti riferiti, tra l'altro, anche all'insegnamento della lingua italiana. La stessa direttiva destina pure venti milioni di euro per iniziative promosse a livello nazionale. Quanto all'undicesimo punto, concernente la promozione di azioni volte a favorire la partecipazione attiva degli studenti immigrati e delle rispettive famiglie, anche attraverso l'attivazione di corsi di lingua italiana nonché di corsi di educazione civica, si ricorda che la suddetta mozione dell'onorevole Cota, approvata dall'Assemblea della Camera il 14 ottobre scorso, si muove già in tale direzione, laddove prevede l'elaborazione di un curricolo formativo essenziale che tenga conto di progetti interculturali

concernente la realizzazione di un'offerta didattica per gli immigrati adulti regolarmente soggiornanti, la suddetta direttiva ministeriale n. 69 del 6 agosto 2008 colloca lo sviluppo dell'istruzione permanente per gli adulti tra gli interventi prioritari da porre in essere, nell'ambito delle collaborazioni istituzionali con le Regioni e gli enti locali. In merito, poi, al tredicesimo punto, si ricorda che la vigente convenzione con la RAI contempla il progetto Italiano «L2», destinato all'alfabetizzazione e alla diffusione della lingua italiana di base per stranieri adulti di nuova residenza

che in modo acritico si sono avvicinati alla lettura delle nostre proposte, perché poi non ci siano equivoci sulle questioni. Leggo e cito testualmente da «la Padania» del 15 ottobre 2008: «Queste classi dunque serviranno ad insegnare la lingua, ma anche ad inserire nel contesto sociale i piccoli alunni». Si faranno cioè delle classi separate, si farà un test d'ingresso, si terranno dei corsi per la lingua italiana e corsi di educazione civica per capire se i bambini sono nelle condizioni di comprendere la nostra Carta costituzionale.

venti minuti. Abbiamo cercato di dirvi quali sono gli strumenti che dovete utilizzare per consentire l'integrazione. Non potete continuare a prendere in giro anche i cittadini padani dicendo che fate le classi ponte, che sono altra cosa sul piano culturale (spregevole), sapendo che non si possono fare. Questo modo di governare

siamo determinati nel votare a favore di tutte e tre le mozioni, quella a prima firma D'Alia, quella a prima firma Giambrone, condivisa dall'intero Gruppo dell'Italia dei Valori, e quella a prima firma Soliani. Abbiamo esposto le ragioni nell'illustrazione della mozione e quindi insistiamo nelle nostre richieste e nell'approvazione delle mozioni stesse.

la Lega Nord, dopo aver recepito tutti gli interventi in sede di discussione generale, intende intervenire in dichiarazione di voto ribadendo il proprio sentire. Quando esponenti della minoranza sostengono che per realizzare un vero processo di integrazione non bastano le leggi ma serve il dialogo e la condivisione tra le culture, hanno ragione. Ma è pur vero che senza la valorizzazione delle proprie certezze identitarie, ogni dialogo è destinato a risolversi nel relativismo presente in ogni forma di multiculturalismo. La Lega Nord afferma che chi possiede la coscienza di sé, dei propri valori identitari e delle proprie radici culturali, possiede anche la capacità di aprirsi agli altri facendo però valere le proprie irrinunciabili ragioni. E sono le ragioni del nostro ordinamento giuridico, della nostra democrazia e del rispetto per la dignità e la libertà di ogni singola persona. Sono ragioni non negoziabili. Solo gli Stati europei che oggi hanno il coraggio di chiedere agli immigrati il rispetto e la condivisione delle regole e delle radici culturali, attraverso una più completa istruzione e formazione ed attraverso la conoscenza adeguata, nel nostro caso, della lingua italiana, sono anche quelli che intendono realmente aiutare i lavoratori stranieri ed i loro figli. Questo è ciò che Lega Nord vuole per la sua gente e per gli stranieri. Non a caso la Lega Nord ha recentemente presentato alla Camera la mozione in cui si chiede al Governo di impegnarsi alla realizzazione delle classi di accoglienza per quegli alunni stranieri che non conoscono la lingua italiana, in deroga al Regolamento di cui al decreto del Presidente della

Disegno di legge che prevede che gli alunni stranieri possano usufruire di corsi di *full immersion* nella lingua italiana dello studio e di percorsi didattici di educazione alla legalità, alla cittadinanza ed alla convivenza civile. Si tratta di un disegno di legge di buon senso. senso. Vi leggo ora un'opinione: «Dare agli studenti la possibilità di imparare prima la lingua in classi costituite appositamente a tale scopo, è non solo il contrario di razzista: è moralmente doveroso. Prima di gridare al lupo contro un presunto governo razzista, sarebbe meglio riflettere bene su quel che è lo stato concreto delle cose. Non riesco davvero a trovare ragioni sostenibili per la totale interdizione, se non attingendo al repertorio della contrarietà ideologica, solo per creare ostacoli all'avversario. L'inserimento brusco in una classe normale, sarebbe esso sì, una forzatura, un'azione che potrebbe sortire lo scoraggiamento dall'impossibilità di padroneggiare le materie di studio». Chi afferma ciò è il responsabile della scuola araba di Milano che certamente non è leghista. La normativa attuale prevede il brusco inserimento in una classe normale generando forzature e scoraggiamento; e le mozioni oggi in discussione auspicano il mantenimento dello *status quo*. Già una volta vi ho chiesto di vedere gli occhi smarriti dei bambini che non capiscono le parole della maestra e dei compagni. Eppure voi oggi insistete chiedendo di lasciare tutto così com'è. Quei dirigenti scolastici, collegi dei docenti, genitori italiani e stranieri che già oggi stanno sperimentando le classi ponte su al Nord, vi guarderebbero sgomenti esclamando: «Ancora!!??» Così come sono rimasta scandalizzata leggendo, qualche settimana fa su un quotidiano, che in una scuola media era stata creata una classe ponte sperimentale inserendovi gli alunni stranieri e quelli portatori di *handicap*. Questi insegnanti hanno davvero calpestato la dignità degli alunni stranieri e dei diversamente abili, ma non hanno mancato di sputare gratuite sentenze contro la Lega Nord dalle righe del quotidiano. La Lega Nord voterà contro le mozioni, perché non vengono incontro alle richieste di un cambiamento di rotta formulate dai territori ad alta immigrazione; perché non ci si è accorti che a fronte di tante sperimentazioni positive di modelli diversi di classe-ponte, si corre il rischio di realizzare delle pericolose devianze tipo quella citata e perciò si rende necessario discutere, confrontarsi e condividere per normare l'esistente; mozioni si chiede la modifica dei contenuti dei programmi scolastici obbligatori, avviando la scuola al multiculturalismo che la gente non vuole. A tal riguardo faccio presente ai senatori Peterlini, Pinzger e Fosson che oggi hanno fatto comprendere ai loro elettori che sono disposti a farli rinunciare all'insegnamento della lingua e della cultura tedesca o francese nelle scuole dei loro territori, per dare spazio all'interscambiabilità delle culture e delle religioni quale mezzo migliore per l'integrazione degli alunni italiani con le culture diverse. Perché è questo ciò che voi state chiedendo al Governo a nome dei vostri elettori. L'attuale minoranza cerca di inculcare ai cittadini italiani, salvo poi accusarli di intolleranza se non vi si adeguano silenziosamente, che sono gli alunni e le famiglie italiane che si devono integrare con gli stranieri. La vera riflessione che la politica deve affrontare non è il nome politicamente corretto da assegnare alle classi ponte e nemmeno se sia il caso di istituirle: tutti sappiamo che sono un'ottima soluzione per imparare l'italiano e le regole. La scelta che la politica deve fare è se si ritiene prioritario inserire a scuola i minori stranieri favorendone l'integrazione attraverso l'apprendimento vero della lingua italiana e delle lingue locali, che sono espressioni delle radici culturali, storiche, giuridiche dei diversi territori e attraverso l'apprendimento e l'assimilazione delle nostre regole di convivenza civile; oppure no. La Lega Nord voterà contro le mozioni perché in realtà non permettono ai minori stranieri la pari opportunità di accesso allo studio e di successo scolastico e perché col solito buonismo chiedono alle famiglie italiane la negoziazione di valori ed identità culturali che per gli elettori della Lega Nord non sono negoziabili. negoziabili. Signor Presidente, per onorare il suo invito a parlare brevemente dovrò tenere nel cuore molte osservazioni, che non sono risposte necessariamente ai colleghi della Lega: non ho sentenze da sputare. Ma ogni volta che parliamo di scuola in quest'Aula ho davvero la sensazione che, siccome siamo stati insegnanti, pensiamo alla scuola di oggi e di ieri e invece questa è la sede in cui si prepara la scuola del futuro. tribuna studenti di un liceo classico che ci ascoltano e mi rammarico che abbiano dovuto sentire che in quest'Aula, invece di pensare che sia la scuola ad integrare, si pensa che sia la scuola che crea

*(PdL)*. Signor Presidente, sottosegretario Pizza, onorevoli colleghi, stiamo parlando oggi di una questione molto importante per questo Paese, che credo sia anche fondamentale per il suo futuro e che vede che vede sicuramente, nella forza degli immigrati, una forza lavoro significativa per l'economia stessa. Ebbene,

Se comprendiamo questo, probabilmente il dibattito andrebbe portato su un'altra sponda, quella della correttezza, senza dietrologie e senza nasconderci dietro articoli della Costituzione che tutti ben conosciamo, come l'articolo 34 o l'articolo 3. Per fare in modo che l'integrazione sia vera e non sia solo un parcheggio che crea problemi, dobbiamo far sì che gli studenti

corretta nelle nostre istituzioni, come giustamente afferma una vostra amministrazione di centrosinistra, che qualcuno poc'anzi ha ricordato; e dovrete anche mettervi d'accordo una volta per tutte tra ciò che affermate in Parlamento

che i figli degli immigrati dovranno presentare domanda di iscrizione alla scuola entro febbraio, i Comuni dovranno comunicare alla Provincia nome, paesi d'origine e lingua madre degli studenti, che non potranno frequentare le lezioni se prima non avranno raggiunto un livello minimo di conoscenza linguistica. Questo dicono il governatore e l'assessore all'istruzione della Provincia di Bolzano,

per età, senza pensare alle loro conoscenze. Faremmo un danno a loro, esclusivamente a loro, e non è un modo per integrarli, ma anzi è un modo chiaro per allontanarli dalla scuola. Vedete, dobbiamo porci un'altra domanda molto semplice: quale scuola vogliamo? Quale istruzione vogliamo? Perché se la scuola è solamente un contenitore che deve dare conoscenze nulle, vuote, cultura zero, allora è la vostra scuola. Noi vogliamo un'altra scuola, che dia cultura e conoscenze, sia ai nostri ragazzi sia, e soprattutto, ai ragazzi stranieri che devono integrarsi, perché noi crediamo fermamente in una vera integrazione.

si legge l'impegno per il Governo a preparare approcci nel settore linguistico integrati con le attività pratiche, differenziando

come giustamente previsto dalle normative del 1998 e del 2002, che danno indicazioni utili sulla funzione dei cosiddetti spazi dotati di strumenti appositamente dedicati, demandando alle scuole e agli enti locali iniziative per la gestione di tali spazi e strumenti mirati all'istituzione di percorsi specifici di alfabetizzazione linguistica. Questi sono gli strumenti che vanno applicati, queste le strade che vanno percorse, e non altre. Ebbene, siamo contrari

Questo è il vero danno, il vero razzismo, non l'altro. Questa è la verità, ed il Paese reale è lontano da voi e dalla vostra politica e lo sta dimostrando tutti i giorni. Oggi voi ancora non ve ne rendete conto,

che gli strumenti saranno posti ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

di impegnare il Governo a «concorrere a definire urgentemente in sede internazionale le competenze per il giudizio nei confronti dei responsabili di atti di pirateria anche in un foro internazionale *ad hoc*», lasciando aperte tutte le possibilità.

ricordare l'importanza degli interessi economici che l'Italia ha in quell'area e degli approvvigionamenti energetici strategici per tutto il sistema europeo,

jihadista che fa riferimento ad Al Qaeda e che si sta sempre più radicando, in particolare, nei Paesi falliti che si trovano allo sfascio, come oggi è la Somalia. Per la sicurezza internazionale, contro il terrorismo e a favore del nostro sistema economico,

L'importante è che rimanga che oggi possiamo sconfiggere il crimine della pirateria non perché abbiamo norme di diritto interno, ma per norme consuetudinarie di diritto internazionale. Il problema è che, pur trovando un'applicazione nella fonte

Governo è stato sfiduciato dal Presidente della Repubblica, ma si è votato di nuovo la fiducia; quindi è una situazione completamente fuori controllo. Sappiamo che queste azioni di pirateria possono finanziare non soltanto la criminalità organizzata di stampo generico, ma anche attività terroristiche. Vi è anche un motivo umanitario, che abbiamo inserito nel dispositivo della mozione. In quel Paese la situazione è drammatica per milioni di persone e, da questo punto di vista, il fatto che ci siano atti di pirateria impedisce anche l'arrivo di aiuti umanitari. Quindi, non è semplicemente un problema che riguarda il mondo altro rispetto alla Somalia.

questa mozione, sia molto importante. Ritengo che sia altrettanto rilevante quanto possono fare le nostre Forze armate. Una nostra nave, il «Durand de la Penne», è rientrata il 12 dicembre con l'ammiraglio Gumiero; mi unisco ai ringraziamenti che sono stati già rivolti per il lavoro Si chiede al Governo di poter continuare questo impegno. Da missione NATO è diventata una missione dell'Unione europea. Il comando è attualmente britannico partecipano la Francia, la Germania, la Grecia, oltre alla Gran Bretagna. Credo sia importante per l'Italia mantenere un impegno, proprio perché se oggi diciamo che vi è un'emergenza - ed è un'emergenza internazionale - non ci possiamo sottrarre a questo problema.

In particolare, su questa spinta è nato l'ordine del giorno a firma Rutelli ed Esposito e su questa spinta sono nate le nostre considerazioni su un'area abbandonata a se stessa negli ultimi vent'anni.

denominata "Atalanta"; a concorrere a definire urgentemente in sede internazionale le competenze per il giudizio nei confronti dei responsabili degli atti di pirateria, con l'obiettivo di individuare uno specifico foro internazionale *ad hoc*.

proposta, da un lato salvaguardi l'attuale giurisdizione e dall'altro dia il forte segnale politico di voler creare una nuova e diversa situazione rispetto all'attuale per quanto riguarda i giudizi sui pirati.

episodio, denunziato dall'avvocato Antonio Fiumefreddo (che, tra l'altro, è il soprintendente del teatro Bellini di Catania, oltre che ben noto penalista)

(che sarebbe stato anche un detenuto operante nell'ambito di una cosca mafiosa e quindi ristretto per motivi riguardanti tale sua compromissione), il quale, accusato da altri più anziani ed autorevoli - per così dire - detenuti, sempre appartenenti alla famiglia mafiosa, di essere un omosessuale per il suo comportamento e per essere dedito alla composizione di versi poetici,

di questo fatto non denunciato dall'ultimo pervenuto e che anzi era stato ripreso nell'ambito di un'intervista rilasciata dal dottor Antonio Ingroia, procuratore della Direzione per sapere se rispondesse al vero e, ove mai così fosse stato, se fossero stati adottati provvedimenti di punizione a carico degli autori di un così efferato delitto e quali misure si fossero adottate per la sicurezza

qualunque sia il detenuto, quali che siano le sue inclinazioni sessuali, financo le ragioni della sua restrizione in carcere, è di tutta evidenza che in un Paese civile, quale ci onoriamo di essere, ove mai un episodio del genere fosse rispondente al vero, è intollerabile che esso resti non accertato, non adeguatamente sanzionato e che non venga assicurata la sicurezza fisica del ristretto, specie in questo contesto. Ebbene, il Ministero si è

ho appreso che il giovane, definito mafioso, comunque poeta, presunto omosessuale e presunta vittima di stupro, si è impiccato. sono turbato da questo episodio, profondamente turbato, perché la vita umana, in qualunque persona

finestra"). Senatore Ceccanti, la Presidenza si farà carico di sollecitare il Ministro perché, alla ripresa dei lavori dopo la pausa delle festività natalizie,

*(PD)*. Signor Presidente, nel mese di ottobre, un po' come è avvenuto questa mattina, il Senato si è trovato ad adottare unanimemente un ordine del giorno, seppure con la non partecipazione al voto della senatrice Poretti e mia, relativamente alla persecuzione dei cristiani. In quella fase, anche se forse un po' meno di oggi, si auspicò un dibattito più ampio, che potesse portare l'Assemblea all'adozione di un documento sicuramente più ragionato e più articolato, possibilmente non degradandolo ad ordine del giorno come, ahimè, è avvenuto oggi,

con l'onorevole Marco Pannella da domani mattina visiterò prima la Cambogia e poi il Vietnam proprio per tentare di acquisire informazioni relativamente a due gruppi gruppi perseguitati: il primo, cristiano protestante, sugli altopiani centrali del Vietnam; il secondo è la Chiesa buddista unificata non riconosciuta dal Governo di Hanoi. La nostra presenza colà è stata ampiamente pubblicizzata anche con le autorità vietnamite, che proprio ieri hanno voluto inviare una delegazione di parlamentari all'Europarlamento a Strasburgo, dove in qualche modo si è minimizzato qualsiasi tipo di persecuzione religiosa ai danni di minoranze etniche o di chiese che non siano formalmente iscritte presso il Ministero degli esteri. Sarà mia cura, una volta rientrato, entro la fine dell'anno, anche fornire un resoconto di missione.

Signor Presidente, l'intervento del senatore Benedetti Valentini mi consente di affrontare un tema che mi ero già ripromesso di sviluppare oggi proprio per porre l'accento su quanto sta accadendo all'interno delle carceri italiane e siciliane in particolare. Le carceri stanno scoppiando, il Sistema sanitario nazionale non ha ancora provveduto - o almeno non dappertutto - ad attuare le disposizioni previste per il passaggio delle competenze della sanità penitenziaria al Sistema sanitario nazionale, il sovraffollamento delle carceri medesime e tutta una serie di fenomeni legati alla carenza di personale di guardia e di assistenza (in particolare di psicologi) stanno purtroppo determinando una condizione estremamente allarmante nelle carceri italiane. Gli episodi a cui ha fatto riferimento poc'anzi il senatore Benedetti Valentini sono uno falso e l'altro vero: il primo, quello che riguarderebbe presunte violenze sessuali subite da un giovane omosessuale e poeta nel carcere di Piazza Lanza di Catania è del tutto destituito di fondamento, non solo perchè io stesso, per altra funzione che esercito, ho potuto accertarlo per l'indagine avviata in tal senso e per le verifiche fatte presso l'infermeria del carcere e presso gli ospedali cittadini,

mai stato avvocato di nessun custodito nelle carceri di Piazza Lanza di Catania avente le caratteristiche del del soggetto che sarebbe stato sottoposto a violenza. Dunque una bufala clamorosa, purtroppo ripresa da molti giornali, alcuni dei quali altrettanto strumentalmente imbeccati. L'altro episodio, quello di due giorni fa, purtroppo è vero: è un episodio di suicidio che deriva da altra violenza e che riguarda altro soggetto, nel presupposto che il primo non esista e questo sì. Un soggetto non omosessuale, che non scrive poesie, che ha subito delle violenze, che è stato trasferito da un carcere all'altro a causa delle violenze subite e che ha più più volte segnalato per iscritto e attraverso i suoi avvocati e che muore suicida, come moltissimi detenuti italiani muoiono suicidi. Purtroppo il dato è in forte aumento, soprattutto perché l'assistenza psicologica garantita dall'amministrazione penitenziaria nelle carceri italiane è assolutamente minima,

è soltanto uno o al massimo due durante la loro detenzione perché esiste una carenza cronica di psicologi nelle carceri. Paradosso aggravato dal fatto che un concorso appena appena completato e quindi già esecutivo non viene sbloccato con la relativa assunzione del personale. Concludo, signor Presidente, chiedendo al Parlamento di attivarsi con gli strumenti previsti dal nostro Regolamento per affrontare un tema delicatissimo, quale quello della istituzione di un Ufficio del garante nazionale dei diritti dei detenuti, che certamente potrebbe servire, non solo collaborando con i garanti già esistenti nel territorio, ma proprio in casi come quelli segnalati dal senatore Benedetti Valentini che destano clamore e confusione e che certamente non valgono a risolvere i problemi gravi delle carceri che, invece, sono purtroppo sempre più crescenti e sempre più allarmanti.

Penso che il Governo potrà riferire sull'insieme di questi episodi, in modo che vi sia questo approfondimento, così come era stato chiesto in un'interrogazione.